Comunico che in data 17 luglio 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la seduta costitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, già prevista per oggi, è rinviata mercoledì 26 luglio 2023, alle ore 14, presso la sede di Palazzo San Macuto. La seduta costitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, già prevista per mercoledì 19 luglio 2023, alle ore 8,30, è rinviata a martedì 25 luglio 2023, alle ore 13, presso la sede di Palazzo San Macuto. La seduta costitutiva della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, già prevista per mercoledì 19 luglio 2023, alle ore 14, è rinviata a mercoledì 26 luglio 2023, alle ore 8,30, presso la sede di Palazzo San Macuto. La Conferenza dei Capigruppo ha rimodulato il calendario della settimana corrente e approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 4 agosto. Nella seduta di oggi si svolgeranno le discussioni generali del decreto-legge sull'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e del disegno di legge sul divieto di produzione di alimenti e mangimi sintetici. Il seguito dell'esame dei due provvedimenti avrà luogo nella seduta di domani, a partire dal disegno di legge sugli elementi sintetici. Gli emendamenti al decreto-legge sull'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea dovranno essere presentati due ore dopo la trasmissione ai Gruppi del testo approvato dalla Commissione. Giovedì 20 luglio sarà discusso il decreto-legge sul settore energetico. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul testo approvato alla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. Seguirà la chiama. Sempre giovedì 20, alle ore 15, avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri delle infrastrutture, della cultura e per la Protezione civile. Martedì 25 luglio, con inizio alle ore 12,30 e senza orario di chiusura, saranno discusse mozioni che dovranno essere segnalate dai Gruppi entro giovedì 20 luglio, alle ore 12. Per ciascuna mozione, dopo l'illustrazione di cinque minuti, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, anch'esse della durata di cinque minuti ciascuna. Mercoledì 26 luglio, alle ore 10, sarà discussa la mozione di sfiducia individuale al Ministro del turismo. Dopo l'illustrazione, ciascun Gruppo potrà intervenire per cinque minuti in discussione generale e per dieci minuti in dichiarazione di voto e seguirà la chiama. Gli orari della seduta di mercoledì 26 luglio terranno conto della cerimonia degli auguri alla stampa parlamentare prevista per le ore 14,30. Il calendario della prossima settimana prevede inoltre la discussione dei disegni di legge sul rendiconto e assestamento e del decreto-legge sugli interventi per gli eventi alluvionali, attualmente alla Camera dei deputati. Il calendario della prima settimana di agosto prevede altresì la discussione del decreto-legge pubblica amministrazione, sport e giubileo, attualmente all'esame della Camera dei deputati, nonché del disegno di legge delega fiscale, approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra di finanza pubblica.

Presidente, intervengo per chiedere al Governo un'informativa urgente del ministro degli affari esteri, Antonio Tajani, su quanto è accaduto a Patrick Zaki oggi in Egitto. Si chiude oggi drammaticamente il primo tempo dell'incubo che lo insegue dal febbraio di tre anni fa, l'incubo di una persecuzione che ha portato questo ragazzo a passare un anno e mezzo in un carcere egiziano e a dormire per terra: una tortura, per poi trovare un sollievo parziale e provvisorio con la liberazione nel dicembre del 2021, restando tuttavia sotto la scure di un giudizio che veniva rinviato di mese in mese, in un'agonia di diritto e libertà. A Patrick era negata la possibilità di viaggiare, di uscire dal suo Paese, che è diventato un carcere; di potersi laureare in presenza nella sua Bologna, com'è successo ancora qualche giorno fa. Oggi la sentenza a tre anni di carcere - saranno quattordici mesi - una mazzata per questo ragazzo, per la sua famiglia e per l'intera comunità internazionale che si è mobilitata in tutti questi anni per la sua liberazione. Due anni fa, Presidente, chiedemmo sia alla Camera dei il conferimento della cittadinanza onoraria per Patrick. Approvammo la mozione, ci portammo a casa le belle parole, ma Patrick è rimasto in Egitto e non è diventato cittadino italiano. Abbiamo chiesto all'attuale Governo di attivarsi per consentire a Zaki di poter viaggiare, come sono riusciti a fare altri attivisti sotto giudizio: nessuna risposta dal Governo; un silenzio che oggi si allunga come un'ombra di fronte all'abuso

le prese in giro, le responsabilità, le menzogne, cosa intende fare oggi il nostro Governo nei confronti del regime egiziano? *(Applausi)*. Venga qui a dircelo. Noi continueremo la nostra mobilitazione al fianco di Patrick, della sua famiglia, dei dissidenti torturati e imprigionati, dell'ansia di libertà di un ragazzo che voleva solo studiare a Bologna. *(Applausi)*.

il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea e della legge europea relativa agli anni di riferimento.

dei caratteri di una Nazione impegnata a migliorare la qualità e la diffusione del lavoro, la salute dei cittadini, il rispetto dell'ambiente, e a sostenere la diversificazione ecologica e la sicurezza energetica, con il Governo Meloni che opera incisivamente nella formazione dei giovani e della scuola. Le soluzioni individuate di concerto con le istituzioni europee hanno in diversi casi rilevanza critica nell'attuazione del mercato unico, nel sostegno della crescita e dell'occupazione, nel creare condizioni più eque di concorrenza e nel riconoscere reciprocità e rispetto al *made in Italy*, alla nostra tecnologia e alla nostra ricerca. un orizzonte vasto quello a cui guarda il Governo Meloni, con soluzioni date a numerose procedure di infrazione aperte e insolute da tempo o in fase di pre-infrazione e in alcuni casi *in fieri*, ma sicuramente agevolmente prevedibili. In tale ottica, la finalità del decreto-legge è quella di ridurre il numero delle procedure di infrazione. Con il disegno di legge in esame si procede a stabilire disposizioni normative che possano portare alla chiusura di circa tra procedure di infrazione e pre-infrazione: una quota molto alta di interventi che dimostra concretamente l'impegno italiano nell'adempimento degli obblighi europei e come l'Italia di oggi sia un *partner* credibile, affidabile e convinto sostenitore del progetto europeo. Abbiamo una visione molto chiara dei rapporti tra gli Stati membri, la loro sovranità e la necessaria dimensione europea, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. È un percorso, quello del processo di adeguamento alla normativa europea, che risponde peraltro a una visione e a un mandato preciso di questo Governo. In Commissione sono stati approvati numerosi emendamenti, con il contributo del Governo, autorevolmente rappresentato dal ministro Fitto, dal ministro Ciriani e dalla sottosegretaria Castiello, che ringrazio in modo particolare per il costante impegno. Tra i molti emendamenti approvati in Commissione, ricordo quelli del Comitato per la legislazione presieduto dal senatore Matera, che ha contribuito a migliorare sostanzialmente il testo proposto dal nostro Esecutivo. Si è discusso molto in Commissione anche sul tema della proponibilità degli emendamenti. Mi permetto di ricordare come lo strumento principale per l'adeguamento degli obblighi europei sia costituito dalla legge n. 234 del 2012, dalla legge europea e dalla legge di delegazione europea, sempre ai sensi della legge n. 234. Ho ritenuto opportuno e necessario circoscrivere la proponibilità degli emendamenti, in linea con quanto prescritto dall'articolo 36 della legge n. 234, ai soli emendamenti che presentassero un contenuto ragionevolmente omogeneo con l'adempimento necessario di un obbligo europeo e presentassero connotati di urgenza. Ringrazio tutte le forze politiche presenti in Commissione per il loro atteggiamento costruttivo, pure in un contesto di confronto anche marcato, su alcuni singoli temi, come ad esempio il tema dell'Ilva. Vorrei anche rilevare il punto relativo al tema, importantissimo per la nostra credibilità europea e per la coerenza con le normative europee e con le politiche europee di finanza pubblica, dell'invarianza della spesa, che talvolta ci obbliga, purtroppo, a non accogliere proposte certamente utili e di assoluto buon senso,

per l'applicazione degli strumenti previsti dalla legge n. 234 riguarda la presentazione alle Camere di due disegni di legge europea e di due disegni di legge di delegazione europea ogni anno. La finalità è quella di snellire l'*iter* di approvazione dei singoli provvedimenti ed evitare l'adozione di provvedimenti di urgenza. Il disegno di legge che discutiamo oggi comprende 38 articoli, che quindi sono un numero considerevolmente maggiore rispetto ai 27 originali. Non li descrivo in dettaglio, perché sono conosciuti dalla documentazione. Andando però rapidamente vorrei ricordare che il primo riguarda una modifica al testo unico bancario, per risolvere il caso EU Pilot-Fisma relativo al recepimento della della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi. L'articolo 1-*bis* è stato introdotto a seguito di un emendamento del Governo in materia di crisi di impresa, in coerenza con i princìpi della direttiva UE 2019/1023. L'articolo 2 prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso, con un'imposta agevolata di registro dal 9 per le persone trasferite all'estero per motivi di lavoro che abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni. L'articolo 3 riguarda la fine della risoluzione della procedura di infrazione per mancato recepimento in materia di revisione legale dei conti delle società. 3-*bis* reca misure di attuazione della direttiva UE 2019/882 sui requisiti di accessibilità a prodotti e servizi per le persone con disabilità. disposizioni volte a risolvere procedure di infrazione nel processo minorile, informando dell'avvenuto arresto o fermo del minore altra idonea persona maggiorenne in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale. reca modifiche all'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali da funzionari internazionali. mira a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea in ordine alla violazione dei principi di libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria. L'articolo delle medie annue di attività di *radon* nell'aria superiori ai livelli di riferimento consentiti dall'Europa. L'articolo 8 prevede l'istituzione di un fondo per la prevenzione e riduzione del *radon* in ambienti chiusi. In Commissione In Commissione politiche dell'Unione europea è stato anche approvato un emendamento del Governo che reca disposizioni in materia di misure e attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Parliamo dell'emendamento Ilva, che è stato proposto dal Governo e adottato dalla Commissione politiche dell'Unione europea. Vi sono poi altri articoli in materia di pratiche che hanno un'influenza pesante sulle condizioni dell'ambiente e della CO2, l'abbruciamento di materiali vegetali. Poi ci sono altri articoli molto importanti nel campo del pubblico impiego, dell'educazione, della scuola, dell'alta formazione musicale e artistica. In Commissione è stato approvato un emendamento trasversale a molti Gruppi, con cui si fissa un'ulteriore disciplina per il reclutamento del personale AFAM per gli anni accademici 2003 e 2024. Si tratta di un tema dibattuto, perché riguarda il *dies a quo* di applicazione di una normativa che agevoli l'inserimento dei docenti precari o temporanei nei ruoli di questi istituti. istituti. C'è poi una serie di disposizioni riguardanti sempre la funzione pubblica. Ma su AFAM vorrei rivolgermi al senatore Lombardo, per gli sforzi effettuati nell'arrivare a una soluzione condivisa tra le forze di maggioranza e di opposizione, in modo da dare un segnale importante di attenzione ai lavoratori che operano, ai docenti e di riflesso anche agli studenti degli istituti di alta formazione artistica e musicale. In Commissione abbiamo portato alcuni correttivi, tra cui il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della partecipazione a procedure selettive. Vi sono molte altre disposizioni. Fra queste vorrei segnalare in particolare l'approvazione di un importante articolo, il 18-*bis*, con un emendamento a prima firma del senatore Malan, che reca modifiche alla disciplina del mandato di arresto europeo in esecuzione della sentenza del 6 giugno 2023, resa su ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale. Tale emendamento è importante perché garantisce l'applicazione di determinate condizioni alle quali il mandato europeo deve uniformarsi per l'Italia nei confronti di cittadini italiani o stranieri, in base a norme e regole ben fissate dalla Costituzione e dalla Convenzione di Strasburgo. Ho citato alcune tra le molte cose che sono contenute in questo disegno di legge legato al precedente decreto-legge in conversione. Vorrei ringraziare tutti per il contributo dato ai lavori e soprattutto esprimere un rinnovato ringraziamento alla rappresentante del Governo, che ha seguito i lavori in Commissione, al ministro Fitto e al ministro Ciriani. *(Applausi)*. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Scurria.

tra i 27 attuali Stati membri dell'Unione europea, che ha più infrazioni, la maglia nera dell'Europa, così come venivamo chiamati a Bruxelles e non solo. Non c'è stato un solo Governo, dai primi anni duemila, che abbia trovato la voglia, il tempo e la capacità di mettere mano a questo aspetto, che colpisce fortemente l'immagine, la reputazione e anche le casse dello Stato italiano. In realtà, c'è stato un Governo che questa azione ha messo in campo: era il 2009 e - guarda un po' il caso -era comunque di centrodestra. Poi nulla di fatto con tutti gli altri Governi, magari super-europeisti, che davano lezioni a tutti su come ci si dovesse comportare con Bruxelles; Governi fatti spesso da partiti che altrettanto spesso criticavano e mettevano in luce, secondo loro, l'inadeguatezza di un possibile Esecutivo di centrodestra, soprattutto se guidato da Fratelli d'Italia.

e certezza del rispetto delle direttive, dei regolamenti e delle regole; serve l'impegno a ripristinare la correttezza istituzionale tra Unione europea e gli Stati membri. quindi a sanare almeno 35 delle infrazioni che gravano su di noi, per continuare a essere protagonisti e credibili a Bruxelles come per tanti altri risultati che stiamo ottenendo: pensare all'incredibile accordo fatto con la Tunisia poco tempo fa dal Governo italiano, che ancora una volta ha trascinato l'Unione europea a diventare protagonista insieme all'Italia stessa nel Mediterraneo, per mettere in evidenza un aspetto che nessuno credeva potesse essere fatto in così poco tempo.

a tutelare intere categorie e territori; c'è il lavoro fatto tra Governo e Parlamento, in taluni casi - voglio sottolinearlo - con la partecipazione attiva dell'opposizione, con cui abbiamo dato una risposta a tanti aspetti. Ne parleranno sicuramente anche altri colleghi dopo di me, ma abbiamo dato una risposta contro la precarizzazione dei docenti; abbiamo scritto parole chiare sui prodotti del tabacco non da fumo senza processo di combustione; abbiamo tutelato insieme i produttori di tabacco e le aziende che lavorano in questo settore; siamo intervenuti sui produttori del settore latte, sul tema degli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, sul mandato di arresto europeo, sull'Ilva. Abbiamo cambiato una parte della nostra Italia. In particolare, sull'Ilva, visto che ovviamente su questo tema non poteva mancare una certa polemica anche da parte dell'opposizione, vorrei ricordare che l'emendamento presentato dal Governo, e che è stato poi approvato ed inserito nell'attuale dispositivo, pone degli elementi molto importanti, perché chiude finalmente una procedura d'infrazione che pende sullo stabilimento Ilva di Taranto dal 2013 alla mancata adozione da parte delle competenti autorità italiane, che non erano quelle che oggi governano il Paese, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento. Con questo emendamento inserito all'interno del dispositivo abbiamo anche eliminato ulteriori procedure d'infrazione relative alla qualità dell'aria, sempre in riferimento a quello stabilimento; abbiamo continuato e proseguiamo nell'attività di modernizzazione e decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto; abbiamo definito i criteri per attuare i progetti di decarbonizzazione. citato emendamento prevede inoltre che tutti gli obblighi previsti in capo al primo acquirente dello stabilimento dovranno essere rispettati anche dai successivi acquirenti, fino a quando non venga accertata la cessazione dei rischi connessi alla produzione in questa maniera. Si tratta, dunque, di un intervento pone in sicurezza tanti aspetti. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma soprattutto vogliamo sottolineare che con il decreto-legge in esame c'è un altro pezzetto di Italia che mettiamo a posto, che rimettiamo negli standard europei. risistemiamo ambiti di lavoro, di categorie e cittadini per poter intervenire, lavorare e vivere meglio. È un altro passo per un'Italia diversa, che si scrolla di dosso pregiudizi e scarsa considerazione internazionale. Avevamo promesso che ci saremmo rimboccati le maniche e avremmo lavorato incessantemente. Questo provvedimento va letto anche in questa direzione: rendere l'Italia un Paese nuovo, credibile e che in Europa rispetta gli impegni, chiedendo però di essere rispettata sulle proprie prerogative e sulle proprie necessità. iscritta a parlare la senatrice Bucalo.

Il decreto è frutto di un costante e costruttivo confronto tenuto in tutti questi mesi dai singoli Ministeri con il servizio della Commissione europea, con l'obiettivo di chiudere otto procedure di infrazione e di prevenire l'apertura di altre dodici nuove entro il prossimo mese di settembre. Il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana risulta essere superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea, con un aumento a partire dal 2018: fatto che ha reso necessario adottare misure urgenti, non solo per ridurre il numero di dette infrazioni, ma anche per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie. Il decreto si compone di 25 articoli, che trattano diverse materie: dalla tutela dei risparmiatori alla tutela dell'imputato minorenne. Importanti sono le previsioni contenute negli articoli 7 e 8, che stabiliscono norme relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e obbligano gli Stati membri dell'Unione a predisporre un piano d'azione per il radon. Io, però, mi voglio soffermare soprattutto sugli articoli 11 e 14, che hanno l'obiettivo di scongiurare il deferimento dell'Italia dinanzi alla Corte di giustizia per la violazione della disciplina sui rapporti di lavoro a tempo determinato, procedura di infrazione famosissima, la 2014/4231, riguardante il personale scolastico e delle istituzioni AFAM. Nello specifico, l'articolo 14 prevede che al personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche messe in ruolo a far data dall'anno scolastico 23-24

per adeguarsi a quella che è la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepita dalla direttiva Tale direttiva si poggia su un principio fondamentale, che è quello della non discriminazione tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato. Infatti, secondo tale principio, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in un modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.

È in quest'ottica che va un ordine del giorno di Fratelli d'Italia a mia firma, che ha proprio l'obiettivo di affrontare il fenomeno del precariato nella scuola, fenomeno che ha raggiunto in Italia dimensioni talmente elevate

anche perché, da articoli di stampa, si apprende che, in merito alla reiterazione dei contratti a tempo determinato nel comparto scuola, la Commissione europea potrebbe avviare presto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano. italiano. Da qui l'opportunità di prevedere e di introdurre una più snella procedura di reclutamento. Questo ordine del giorno - è

prevedere e quindi a mettere a regime questa forma di reclutamento straordinario dalle cosiddette famose GPS sui posti comuni e di sostegno,

al fine di accertare la compatibilità di questa riforma del reclutamento con quella prevista dal PNRR, perché sappiamo tutti che il PNRR ha introdotto un'altra riforma del reclutamento volta a garantire 70.000 docenti entro il 2024. Quindi, ancora una volta, ringrazio il Governo per aver accolto il mio ordine del giorno e mi soffermo su un altro articolo molto importante che prevede, per il personale docente tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM, il diritto al riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo del servizio pre-ruolo in servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici. Qui tutto nasce veramente da un piccolo cavillo, perché

Con la legge n. 508, però, non si è previsto nulla sul servizio pre-ruolo e, quindi, è stata applicata, anche se c'era una disciplina diversa, la disciplina precedente. Da qui la necessità di prevedere questo passaggio,

per venire incontro alle istanze degli interessati, perché le istituzioni AFAM potranno indire delle procedure di reclutamento straordinario per risolvere l'annoso problema del precariato;

di andare incontro a un contenzioso. In conclusione, signor Presidente, questo decreto - come ho già detto - ha l'obiettivo di agevolare la chiusura delle procedure di infrazione e dei casi di pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Si tratta di una misura cui da tempo l'Italia non faceva ricorso, esponendosi a richiami e sanzioni. Ancora una volta il Governo Meloni dimostra di essere un Esecutivo del fare e del saper

fatto di essere arrivati a un ammontare di sanzioni di circa un miliardo di euro può essere considerato certamente un buon motivo per intervenire in questa materia anche attraverso un decreto-legge. La necessità è quella di evitarne altre ancora. Quest'anno, dunque, ai tradizionali strumenti normativi previsti dalla riforma delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, se ne unisce uno immediato e immediatamente vigente: un decreto-legge al quale l'esame in Commissione politiche europee ha poi aggiunto ulteriori temi che vanno a meglio precisare il quadro nazionale all'interno di quello europeo. Il tema reale era quello di ridurre il numero di infrazioni, così costoso per le nostre casse e, al tempo stesso, uniformare il nostro diritto a quello comunitario. La media europea è di 66 infrazioni rispetto alle oltre 80 pendenti nei confronti dell'Italia. Così facendo, riusciremo ora a chiuderne circa quattro su dieci, portandoci persino al di sotto della media europea. In generale va notato che il numero medio europeo così alto di infrazioni ci consegna il senso della difficoltà di recepire *in toto* e nei tempi richiesti una normativa europea che è in continuo divenire, in progressiva evoluzione e che tocca ormai ogni aspetto della nostra vita. vita. Condividiamo dunque la necessità e il contenuto del decreto, posto che attraverso di esso è stato possibile anche adottare interventi normativi per fronteggiare alcuni ulteriori obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Pertanto, da una parte evitiamo procedure di infrazione o eventuali sentenze di condanna; dall'altra, ci poniamo in linea con il resto dei Paesi europei, per un altro verso ancora abbiamo persino anticipato la legge di delegazione europea, evitando le modifiche o le abrogazioni delle disposizioni statali italiane non giudicate conformi a quelle europee. un'azione puntuale del Governo, cui hanno contribuito anche i Ministri di Forza Italia per le importanti parti di rispettiva competenza.

Signora Presidente, discutiamo oggi la conversione dell'ennesimo decreto-legge del Governo Meloni.

Questi decreti-legge, invece, non servono per alleviare le sofferenze del Paese o per aiutare i cittadini e le imprese ad affrontare l'attuale momento di emergenza.

solo, questi decreti servono, con un uso strumentale, per andare a togliere e distruggere quelle misure che erano state approvate per favorire i cittadini e le imprese, come il superbonus al 110 per cento, Transizione 4.0 e tante altre misure. Detto questo, entrando nel dettaglio del provvedimento, ho sentito alcuni componenti della maggioranza applaudire il Governo per aver introdotto l'emendamento sulla questione Ilva. È come se la questione Ilva si potesse risolvere esclusivamente con un emendamento buttato lì per caso nell'ultimo giorno di discussione in Commissione e poi portato in Aula per la sua approvazione.

norma salva-Ilva, che di «salva» non ha esattamente nulla. Signora Presidente, volevo evidenziare che questo Governo ha anche un altro *record*: in pochi mesi, quasi nove mesi, è la terza volta che interviene sulla questione Ilva. È intervenuto con il prestito da 680 milioni a favore della continuità produttiva, senza in cambio garanzie sulla restituzione di questi soldi pubblici, ed è intervenuto recentemente anche sulla reintroduzione dello scudo penale. Oggi, su quest'ultimo tema, lo scudo penale, il Governo interviene con questo decreto-legge, che non c'entra nulla con l'infrazione, e addirittura amplia questo diritto ad uccidere (perché è un vero e proprio diritto a uccidere a uccidere che noi andiamo ad estendere), questa volta non solo con riferimento all'attuale continuità produttiva (lo scudo penale si applica a tutta la *governance* attuale), ma addirittura estendendolo al dopo decarbonizzazione.

non sta a significare nulla e non ha alcuna giustificazione. Signora Presidente, ci saremmo aspettati altro in questo provvedimento, dato che si parla di infrazione e le infrazioni europee sono state diverse (nel 2012, 2013, 2015 e tante altre) e hanno riguardato due aspetti importanti, l'impatto ambientale e la qualità dell'aria e quindi, di conseguenza, i limiti degli inquinanti. Con riferimento a questi due aspetti, che sono l'oggetto dell'infrazione, nell'emendamento presentato dal Governo, quello che voi state approvando in questo provvedimento, non c'è nulla che dia soluzione a queste due problematiche. Questo è il tema, per cui vi invito veramente a rispondere a questa domanda: come andiamo a risolvere il problema dell'impatto ambientale e della qualità dell'aria? Noi ci saremmo aspettati altro e per questo abbiamo presentato degli emendamenti in tal senso. Per quanto riguarda l'impatto ambientale si può risolvere in due modi: la chiusura delle fonti inquinanti innanzitutto e, successivamente, se dobbiamo andare a finanziare un processo di decarbonizzazione, questo dovrebbe avvenire in un momento successivo. Però, con riferimento al progetto di decarbonizzazione, cari colleghi, noi avevamo già un progetto di decarbonizzazione che era inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ce lo siamo dimenticati forse. In quel Piano abbiamo anche destinato 1,2 miliardi al processo di decarbonizzazione Ilva. Tutto questo adesso viene completamente cancellato e ciò dimostra, per l'ennesima volta, l'incapacità del Governo di dare soluzione al problema Ilva e ai problemi del Paese.

Quei livelli sono stati ritenuti da diversi studi scientifici, ma anche dall'OCSE e dalla citata direttiva sulla qualità dell'aria, eccessivamente elevati rispetto alla tolleranza umana. Su questo provvedimento, dato che si parlava di infrazione della qualità dell'aria, ci saremmo aspettati anche un intervento del Governo volto a ridurre i limiti degli inquinanti del suddetto decreto legislativo, ma tutto ciò non è accaduto.

l'autorizzazione integrata ambientale, quindi a dare approvazione alla richiesta di AIA. In quella autorizzazione integrata ambientale che è stata richiesta e che il Governo andrà ad approvare

i cinque altiforni oggi in parte spenti, ma si chiede anche l'autorizzazione ad aumentare la produzione a carbone, senza inserire tutele ambientali e sanitarie. La cosa più assurda è che con l'altoforno 2 (Afo2) si chiede di poter bruciare oltre 60.000 tonnellate di plastica, quindi si autorizza a istituire un vero e proprio inceneritore. Per tutti

con gli enti territoriali e con le parti sociali *(Applausi)*, condanna i 4.000 lavoratori che oggi sono in cassa integrazione alla precarietà e condanna all'incertezza tutte le imprese dell'indotto che già hanno subìto perdite per oltre 300 milioni a seguito

la legge di delegazione europea, come qualcuno può immaginare conoscendo anche minimamente come la penso, non è esattamente uno dei momenti che ritengo più alti nella produzione legislativa delle nostre Camere. Ciò perché una legge che va a sanare delle procedure di infrazione sulla nostra attività legislativa

il fatto che non si possa procedere, le procedure di infrazione e così via. Va bene che, con questo rito che ogni anno si compie, in questo caso stiamo parlando di cose che oggettivamente sono di buon senso e che probabilmente sarebbero state in ogni caso recepite nella normale produzione legislativa del Paese. Ma vi posso assicurare che, il primo anno del mio mandato come parlamentare, veder adeguare la legislazione sugli sfalci delle siepi (perché questo era quello che mi era stato presentato nella prima legge di delegazione europea su cui ho avuto modo di

di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni». Questo era stato stabilito dai padri costituenti per l'adesione all'ONU e per l'adesione agli organismi internazionali tendenti alla pace. Non mi risulta che i padri costituenti abbiano mai pensato che le Camere avrebbero dovuto mettersi a legiferare per adeguare gli sfalci delle siepi, rispetto a quello che era stato deciso da qualcuno in Germania, in Polonia o similari, anche perché abbiamo visto e vediamo tutti che le legislazioni europee vengono sistemate in modo chirurgico per non non disturbare mai chi rappresenta in questo momento, ma perennemente, la maggioranza relativa, non perché sono più bravi, ma perché sono di più, vale a dire i tedeschi e i Paesi che fanno loro da satellite. Per cui noi, purtroppo, ci troviamo costantemente a dover adeguare la nostra legislazione su cose che magari non hanno particolare senso. In questo caso, fortunatamente, invece questa legge recepisce, come ho detto, delle questioni che sono quasi sempre di buonsenso devo dire che serve anche per trasmettere a chi ci sta guardando l'utilità della nuova maggioranza di Governo. Basta infatti vedere gli emendamenti che erano stati presentati al per capire come sarebbe stata questa normativa di adeguamento dell'ordinamento alla legislazione europea, se ci fosse stata ancora la maggioranza del PD e del MoVimento 5 Stelle. Cito un emendamento, colleghi, perché almeno così capite che pericolo abbiamo sventato,

carreggiate da una parte e dall'altra, «non può superare il limite di velocità di 50 chilometri all'ora, mentre per le strade (...) locali, tale limite non può superare i 20, massimo 30 chilometri orari». Vi giuro: è scritto proprio così. Cioè, in un emendamento si scrive che non si possono superare i 20, massimo 30

i rischi che fortunatamente abbiamo sventato e che gli italiani hanno sventato con il loro voto, mettendo in minoranza il PD e il MoVimento 5 Stelle, perché altrimenti, a quest'ora, oggi, saremmo qui a dire che si deve andare a 20

cittadini, di fronte all'ideologia *green* che fortunatamente spero abbia i giorni contati. Si spera che alle prossime elezioni europee si metta fine a certe follie che portano alla casa *green*, all'auto *green* e a tutto *green*, che sappiamo benissimo non significa dire che si vuole bene alla natura e che si vuole bene al clima (questo lo vogliamo tutti), ma significa aggravi di costi per i cittadini per cose non utili e in certi casi ideologiche o addirittura dannose.

mantenendo tutta l'occupazione, allora avrebbero potuto tranquillamente farlo prima. Purtroppo invece le cose non sono così semplici e basta governare per rendersi conto che non bastano le parole (mettiamola così). Noi si fa quello che si può, con quello che abbiamo trovato. a parlare la senatrice Rojc. il decreto-legge che ci accingiamo a discutere e a votare è assolutamente inadeguato rispetto all'obiettivo che dovrebbe raggiungere. Esso contiene norme (decisamente troppe) disparate e frastagliate. È chiaro che il Governo vuole usare un decreto infrazioni come grimaldello per ottenere determinati risultati. In Commissione è stata spesso preclusa una discussione vera e approfondita sugli articoli, alcuni anche importantissimi. all'emendamento sull'Ilva, che pone una chiara definizione su come di fatto il ministro Fitto voglia accentrare a Palazzo Chigi tutte Non si vuole dunque la decarbonizzazione dell'Ilva dell'Ilva a Taranto, non ci si cura della salute delle persone, non si pensa a chi verrà dopo di noi e al disastro che questa città, così importante per il Mezzogiorno e non solo, dovrà affrontare in futuro. Un decreto che nasce dalla volontà, proclamata dalla maggioranza, di portare le infrazioni da più di 80 alla media europea di poco più di 60, ma che in realtà si è trasformato in una specie di *omnibus* in cui inserire anche norme decisioni non sempre con finalità chiare, che anzi a volte porteranno a incorrere in nuove infrazioni da parte dell'Europa. Noi abbiamo lavorato per il Paese, proponendo emendamenti corretti e lineari, nati dall'ascolto delle categorie e dei cittadini. Noi vogliamo essere europei e concorrere al benessere dell'Europa rispettandone le regole, che non sono regole non imposte, come spesso si vuole far pensare da parte delle forze della maggioranza, ma condivise con gli altri Paesi in Europa. Non si è voluto normare molte cose; le proposte delle opposizioni sono state respinte a prescindere, tranne rarissime eccezioni. Non si è voluto difendere proposte che normavano, per esempio, il potenziamento del personale dei Vigili del fuoco o sostenere i nostri emendamenti (nostri) sul personale scolastico; e molto, molto altro ancora. Bisognerà riflettere attentamente su quale sia il ruolo che vogliamo avere in Europa. Spesso siete stati pronti a fare la voce grossa in casa, per poi divenire miti europeisti convinti con i Paesi con cui interloquite altrove. L'Italia è stata criticata criticata e sanzionata. Non siamo evidentemente più in grado di ricoprire quel ruolo che spetta ai Paesi fondatori dell'Europa. Spero che, ridiscutendo gli articoli di questo decreto, qualcuno tra i banchi della maggioranza trovi il coraggio di ripensarci.

urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" Questo provvedimento merita un'analisi dettagliata, considerando l'importanza delle questioni affrontate e l'impatto che esse hanno sul nostro Paese e sulla nostra posizione all'interno dell'Unione europea. innanzitutto, come tutti sappiamo, l'appartenenza all'Unione europea comporta l'assunzione di obblighi nei confronti degli Stati membri; obblighi che derivano da atti comunitari come le direttive, i regolamenti e le decisioni, che devono essere recepiti ed attuati nel nostro ordinamento giuridico. Il decreto-legge in questione si pone l'obiettivo di garantire almeno in parte l'adempimento di tali obblighi, fornendo gli strumenti necessari per l'attuazione delle norme europee nel nostro Paese. In pratica, questo provvedimento è composto di norme con le quali il Governo italiano mira al recepimento delle direttive europee nell'ordinamento italiano, affronta le procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dell'Italia e tende a prevenire future procedure di infrazione attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il provvedimento è volto, pertanto, a favorire la riduzione del numero complessivo delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione nei confronti del nostro Paese, che fino all'emanazione di questo decreto-legge era superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea. Venerdì scorso, il 14 luglio, la Commissione ha adottato le decisioni mensili e l'Italia ha avuto l'archiviazione di una procedura (quindi attualmente sono 81). Attraverso disposizioni volte ad agevolare l'archiviazione di otto procedure di infrazione, otto casi di pre-infrazione, un caso di aiuto di Stato e cinque adeguamenti normativi, il decreto-legge n. 69 del 2023 intende accelerare la risoluzione delle infrazioni a carico dell'Italia e prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea. Inoltre, il lavoro della 4a Commissione, presieduta dal presidente Terzi di Sant'Agata, unitamente agli emendamenti del Governo, ha permesso di eliminare almeno ulteriori dieci infrazioni, tra le quali quella pendente per l'Ilva di Taranto, di cui tanto si è parlato in quest'Aula. Si tratta di una scelta politica di grande lungimiranza, dal momento che, una volta raggiunto lo stadio della condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie, può essere molto difficile per uno Stato porre fine porre fine alla violazione del diritto dell'Unione europea, perché molte cose poi non dipendono più dal Governo centrale, con un notevole aggravio per il bilancio dello Stato, che aumenta nel tempo a causa delle penalità di mora.

La riduzione delle infrazioni perseguita dal provvedimento in esame appare significativa sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo. Sotto il profilo quantitativo, le 81 procedure attualmente pendenti saranno ridotte, anche grazie alle disposizioni aggiuntive nella fase di conversione del decreto-legge, di più del 10 per cento: ne elimineremo più di 30, avvicinando quindi l'Italia ai livelli degli Stati membri comparabili, quali la Germania e la Francia.

che il decreto-legge intende sanare sono state evidenziate come particolarmente sensibili dalla Commissione europea nel rapporto annuale pubblicato il 14 luglio. Il Comitato per la legislazione che ho l'onore di presiedere ha presentato alcune proposte emendative per il miglioramento della qualità del testo con riguardo ai profili della semplicità, della chiarezza e proprietà della formulazione. Con le modifiche apportate in sede di conversione, in particolare agli articoli 5, 11, 14 e 23, sono stati specificati riferimenti normativi inesatti o incompleti, sono state corrette alcune imprecisioni relative alla decorrenza delle entrate in vigore di singole disposizioni e sono state perfezionate alcune espressioni improprie che avrebbero potuto generare ambiguità interpretative. Come già evidenziato dal Comitato, è essenziale un rafforzamento della programmazione legislativa rispetto all'esigenza di conformare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, così da limitare il ricorso allo strumento della decretazione di urgenza. Però questa volta è stato necessario, perché è proprio grazie a questa scelta del Governo di adottare disposizioni immediatamente efficaci con il decreto-legge di cui discutiamo che sarà possibile accelerare la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia. Promuovere una maggiore cooperazione tra le istituzioni italiane e l'Unione europea, come previsto dal decreto, deve essere l'obiettivo comune da raggiungere. Quando c'è stato e c'è da discutere, negoziare o battagliare in Unione europea con la Commissione nell'interesse nazionale italiano non ci siamo mai tirati indietro. Questo Governo non si è mai tirato indietro e mai lo farà. Ma quando l'interesse nazionale si persegue cooperando tra le istituzioni è nostro dovere farlo, così come fa il presidente Meloni. Non si tratta di essere miti, ma di essere responsabili. È importante sottolineare che il decreto-legge proposto dal ministro Fitto e approvato dal Governo evidenzia l'assunzione di responsabilità dell'Italia nei confronti degli obblighi comunitari e la volontà di mantenere una posizione di rilevanza nell'Unione europea. La pronta e corretta attuazione degli obblighi europei agevola il dialogo con la Commissione ed allontana ogni dubbio, anche il più pretestuoso, sull'affidabilità del nostro Paese. L'approvazione del decreto-legge, quindi, potrà offrire ulteriori strumenti per la tutela politica ed istituzionale degli interessi nazionali, anche in sede europea. L'adempimento degli obblighi europei è un indice di affidabilità della Nazione che aumenta la nostra credibilità ed il nostro peso specifico anche nelle trattative sui grandi *dossier* aperti con la Commissione europea. Penso alla condivisione di Bruxelles degli ultimi giorni sulla proposta di istituire un'unica grande zona ZES per il Sud Italia. Penso alla cosiddetta decontribuzione Sud, che, unitamente alla ZES, aiuterà e permetterà al Meridione d'Italia di iniziare a mettere in moto la propria economia. Infine, penso all'ultima missione del nostro Presidente del Consiglio, onorevole Meloni, in Tunisia che, di fatto, ha portato a casa un primo risultato importante per arginare i flussi migratori in maniera seria e strutturale. In conclusione, signor Presidente, credo che il Governo e poi la Commissione di merito abbiano elaborato una risposta tempestiva e responsabile alle esigenze di attuazione degli obblighi comunitari e di risoluzione delle procedure di infrazione. L'Italia dimostra così la sua volontà di essere un membro responsabile dell'Unione europea, rispettando gli obblighi comuni e lavorando per il benessere dei suoi cittadini. Questo impegno dimostra la determinazione del nostro Governo nel rispettare le regole condivise, per contribuire alla stabilità e all'efficienza della nostra nazione, che rafforza la propria credibilità e reputazione internazionale. Andiamo finalmente a testa alta anche in Europa, non più proni, ma grandi tra i grandi. Grazie, presidente Meloni.

di aver fornito delle osservazioni, sicuramente utili, che continueranno in prosieguo, anche per quanto riguarda l'attività di preparazione delle prossime leggi di delegazione europea e leggi europee.

nei quali il principio di sussidiarietà sulla sovraordinazione della normativa europea rispetto a quella italiana è stato fatto valere dai Governi precedenti per tanti anni. Sono stati prodotti, infatti, regolamenti e direttive

dire che tutte queste norme sovraordinate sono irrilevanti perché riguardano temi sui quali si sono prodotte le procedure di infrazione sulle quali questo provvedimento agisce.

di PM10 e PM5. Quindi si tratta di interventi economici pluriennali che il Governo dispone per affrontare questi temi; riguardano misure ordinamentali nel pubblico impiego - ne hanno parlato i colleghi

questione Ilva, che è stata fatta oggetto negli anni di una serie di procedure di contravvenzione nei nostri confronti. Il provvedimento adotta delle misure di decarbonizzazione, di *governance* e di attuazione. Naturalmente non è un miracolo; sappiamo che la situazione dell'Ilva è stata prodotta da gestioni molto discutibili e da questioni che hanno avuto rilevanza penale

in queste misure di adeguamento alle normative europee, quindi di soluzione delle procedure di infrazione, è stato oggetto di più

che l'apertura alla *governance* - a pensar male si fa peccato come si diceva un tempo, quindi non penso male assolutamente - aprisse anche a ipotesi di inserimento in un complesso industriale strategico di primaria importanza a livello europeo e a livello globale, da parte, magari, di gruppi di controllo di investimenti o di interferenze estere provenienti da Paesi che non sono particolarmente benefici per la nostra economia e la nostra sovranità. Quindi, questi sono alcuni aspetti. Per quanto riguarda

devo notare che vi sono state, nel tentativo di mantenere una omogeneità ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 che ho citato all'inizio, delle insistenze per inserire in questa serie di misure di risposta alle procedure di infrazione anche delle cose che non c'entravano assolutamente niente. Mi sono visto arrivare decine di pagine di emendamenti su temi che nulla avevano a che vedere sulle procedure di infrazione e ho creduto infatti che fossero improponibili. venire a contestare ancora la coerenza e l'impianto del lavoro che abbiamo fatto, che abbiamo portato avanti. Certo, non devo essere io a fare l'avvocato

Come ho già avuto modo di sottolineare anche in quest'Aula - e non mi stancherò mai di ripetere - in una visione effettivamente e proattivamente integrata *one health*, che fin qui è stata poco applicata, dobbiamo imparare dagli errori del passato (anche il «Corriere della sera» oggi apre: «Un errore ignorare il passato») e investire quindi in governo dei rischi, agendo in prevenzione predittiva e in precauzione, che, giusta la *ratio* dell'articolo 7 del regolamento europeo n. 178 del 28 gennaio 2002, se opportunamente declinato in chiave evolutiva, previene il verificarsi di danni nella situazione di incertezza nel medio e lungo periodo sui rischi o financo nella mancata consapevolezza di possibili eventi avversi per la salute e la sicurezza, soprattutto per la salute. Vi faccio un esempio che è di questi giorni, vale a dire che il comitato dei 25 esperti internazionali dell'FDA ha determinato che l'aspartame è un possibile cancerogeno dopo quarant'anni che è in commercio. Questo dovrebbe farci riflettere, perché nella scienza - cito quasi letteralmente, non lo dico io, ma lo dicono professori qualificati - ci sono cose che sappiamo di sapere bene, altre che sappiamo di conoscere approssimativamente, altre ancora che sappiamo di non conoscere e, infine, ce ne sono moltissime che non sappiamo che esistano. Cito ancora dai documenti a nostre mani, perché ne sono rimasta molto colpita: negli ultimi tre casi, il terzo incluso solo per via ipotetica, se vi sono in gioco salute umana, sicurezza personale e sicurezza ambientale, è ragionevole adottare il cosiddetto principio di precauzione - e noi condividiamo principio che è alla base dell'articolato in esame, ma che dovrebbe ispirare in modo assolutamente incisivo l'azione del legislatore e del programmatore in tutti gli interventi, non solo ordinamentali, sul versante della sicurezza, sancendosi che anche per tecnologie, materiali e prodotti in generale, dunque non solo per alimenti che sembrano molto promettenti, si debbano fare delle istruttorie preventive e precauzionali molto approfondite sulla garanzia di salubrità diretta e indiretta, affinché ciò che oggi pare interessante, anche solo per moda o per tendenza, non si dimostri in futuro a incidenza di rischio per la salute e l'ambiente, soprattutto per la salute. Ricordavo, in proposito, che dobbiamo imparare a vedere nelle nuove tecnologie l'opportunità per cambiare paradigma rispetto agli errori del passato, ma, proprio perché dobbiamo farlo e perché di nuovi prodotti e di nuove tecnologie di processo trattasi, dobbiamo far sì che già dalla preserie, destinata a pochissimi e a costi elevatissimi, sia prevista una maggiore attenzione a tutti i rischi, endogeni ed esogeni, a tutela della salute individuale e collettiva, non solo nella produzione, ma soprattutto nell'utilizzo. Per essere ancora più inequivoca, la visione normativa che ci ispira è di non permettere - e non solo per gli alimenti artificiali, ma anche per componenti della mangimistica - che possa entrare sul mercato un nuovo prodotto se non vi è un oggettivizzata e documentata evidenza scientifica di prevenzione di ogni possibile rischio. Mi rendo conto che gli scienziati sono oltremodo orgogliosi di essere riusciti ad ottenere carne artificiale, ma il nostro ruolo di legislatori ci impone la massima cautela, posto che il produttore dovrebbe dimostrare non solo di avere a cuore la sicurezza degli addetti che lo realizzano, ma soprattutto la salute di chi lo andrà a utilizzare. Inoltre, un'altra riflessione endoistruttoria che mi ha oltremodo colpito è che, poiché non sapere se un evento, nel caso di specie l'ingestione di cibi artificiali, è nocivo non equivale a sapere che lo stesso non è nocivo, il superamento del principio di precauzione pretende logicamente che si producano prove positive sull'innocuità del fenomeno indagato *ex ante*, mentre non sono valide prove mancanti sulla sua eventuale nocività, quali quelle ad oggi disponibili per questa tipologia di prodotti. In altre parole, se vi è un potenziale pericolo o evento nocivo di cui non conosciamo il rischio, vale a dire la frequenza degli esiti conseguenti negativi all'esposizione allo stesso, è meglio tenerlo sotto controllo per un lungo periodo di tempo, fino all'accumulo di casistiche significative, sia sulla natura del rischio che sui suoi effetti in una popolazione utilizzatrice. Quindi, l'enunciazione dei pericoli potenziali (prima fase della procedura di analisi e gestione del rischio), in assenza di dati statistico-epidemiologici robusti circa la sua incidenza nella popolazione esposta e consumatrice per almeno dieci anni osservati, impone l'assunzione del principio di precauzione preventivo e proattivo, talché l'onere della prova, volta a dimostrare l'innocuità del fenomeno o la sua rilevanza, data la bassa incidenza, è a carico di chi propone un prodotto o un processo potenzialmente dannosi per i cittadini e per l'ambiente. L'ho fatta un po' lunga, perché non è sempre detto che essere gli unici che pensano una cosa fa sì che sia quella sbagliata: Galileo insegna. È da queste premesse logico-tecnico-giuridiche che discende la concretezza dell'articolato in esame, sicuramente suscettibile di *upgrade* migliorativi che abbiamo immaginato di proporvi in chiave di armonizzazione e coordinamento emendamentale, ovvero rinviando ad un momento successivo, con un'attenta valutazione degli ordini del giorno presentati, in particolare anche per alcuni accorgimenti di carattere terminologico, considerato l'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del regolamento 2283 del 25 novembre 2015 in punto di alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati. Difatti, non vi è neppure univocità lessicale, posto l'impiego di ben 23 diverse denominazioni per questo tipo di prodotti, il che potrebbe suggerire di optare per qualificarli alimenti artificiali e mangimi artificiali per le motivazioni tecniche ampiamente sviluppate nelle documentazioni istruttorie a vostre mani. Non meno degni di nota possono essere miglioramenti e correzioni evolutive di carattere procedurale, per esempio sul coordinamento dei controlli, di garanzia di qualità e di certificazione dei campioni analitici, nonché per la piena armonizzazione dell'approvanda disciplina nazionale con la normativa europea: un esempio per tutti, in tema di cessioni e di acquisti intercomunitari, come pure sul versante dell'impianto sanzionatorio e di alcuni affinamenti utili per una maggiore incisività e coerenza applicativa, come peraltro emersi ai fini di una valutazione di opportunità nel ciclo di audizioni svolte, avendo ben presente, senza atteggiamenti fideistici, non solo la posizione del Governo e di questa maggioranza sul tema, ma il recente *report* FAO di quest'anno, che prende in esame i pericoli potenzialmente connessi con la produzione di carne colturale e li individua lungo tutto la filiera, pur non concludendo in modo risolutivo. Ciò infatti non toglie che vi siano possibili autorizzazioni per gli enti di ricerca - che anzi andiamo a incoraggiare - finalizzati ad approfondire, sviscerare e fugare i dubbi residui, perché anche la FAO ne elenca ben 53 dico 53 - e di questo si tiene conto nell'articolo 2 del disegno di legge in approvazione, considerato il definito ambito oggettivo non escludente, a comprova di non essere in linea in linea di principio - come nello spirito dell'iniziativa legislativa *de quo* - di ostacolo alcuno allo sviluppo scientifico. In altre parole, noi non siamo parte della corporazione dei maniscalchi che era contro l'avvento dell'automobile pur di continuare a ferrare i cavalli. Lo ripeto: pur essendo molto a favore dell'innovazione e della scienza, dobbiamo evitare per quanto possibile incidenti correlati e i potenziali rischi di nocumento connessi e conseguenti, senza ideologie e pregiudiziali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, quello che ci accingiamo a discutere oggi - consentitemi di ringraziare tutta la Commissione agricoltura e in particolare il presidente De Carlo per l'eccellente lavoro svolto un provvedimento richiesto da almeno 1,2 milioni italiani, coloro che hanno firmato una petizione promossa da un'importante organizzazione di categoria, oltre che da numerosi consigli comunali e da quasi tutte le Regioni italiane. quindi definirlo più un provvedimento di iniziativa popolare, che il Governo ha interpretato in maniera eccellente; iniziativa che riflette un sentimento diffuso in tutti noi. Oltre il 72 per cento dei cittadini italiani, difatti, non solo si disgusta di fronte all'idea di dover consumare questa cosiddetta carne coltivata, ma ritiene questa innovazione, di cui peraltro apparentemente non si capisce il bisogno, una minaccia per la tradizione culinaria e il patrimonio gastronomico nazionale. Solo il 18 per cento si dimostra disposto a provarla, mentre il restante 10 per cento è ancora indeciso, richiedendo ulteriori informazioni prima di assumere una decisione. Questa netta opposizione al cibo sintetico è la testimonianza della profonda connessione emotiva e culturale che gli italiani hanno con il cibo. La cucina italiana è radicata nella nostra identità e nei valori della nostra società e i prodotti locali e genuini hanno sempre avuto un ruolo centrale nelle nostre tradizioni. La questione va però ben oltre la semplice preferenza culinaria: il cibo sintetico solleva interrogativi etici e ambientali. Siamo chiari su un punto: questa trovata del cibo sintetico viene proposta come unica alternativa all'inquinamento che produce la zootecnia. È noto che il nostro settore agroalimentare, in particolare quello zootecnico, è sempre più strutturato sulla sostenibilità e sul mantenimento della biodiversità. I nostri allevamenti, sia con le norme relative al benessere animale sia con gli strumenti della zootecnia di precisione, seguono ormai schemi e protocolli finalizzati a minimizzare l'impatto negativo sull'ambiente. Lo dico perché conosco come funziona un'azienda zootecnica. Conosco i sacrifici degli allevatori, me compresa, e vi garantisco che lo facciamo perché ci crediamo, non perché ce lo chiede la politica o perché ce lo impongono le norme. Ogni sforzo e ogni impegno affinché la nostra attività sia sempre più ecosostenibile li compiamo perché ce lo chiede la gente e perché da sempre ci prendiamo cura dei nostri territori, con tanto rispetto e anche con tanto amore. Secondo recenti stime, l'impatto di questa cosiddetta carne sintetica è dalle quattro alle 25 volte superiore rispetto a quello di un prodotto tradizionale proveniente da un allevamento. Mi chiedo: forse ce la proponete per l'esigenza di sfamare una popolazione mondiale in crescita? In realtà, per produrre 44 milioni di tonnellate di cosiddetta carne sintetica, al 2030, così come richiesto dalla domanda globale, si produrrebbero oltre 300 milioni di tonnellate di CO2, contro i 150 milioni di tonnellate che sarebbero prodotti dai nostri allevamenti. La parte ancor più preoccupante, però, è che il meccanismo di produzione è estremamente complesso e le cellule staminali vengono allevate con l'uso di ormoni, che ormai nella nostra produzione zootecnica sono vietati, e anche con una massiccia dose di antibiotici, a fronte di quell'enorme sforzo fatto dagli allevatori per ridurne l'uso, ad ogni vantaggio e per la tutela dei nostri cittadini e dei nostri consumatori, non certo a miglioramento della redditività dell'allevamento. Dico questo per evidenziare che il processo di autorizzazione per l'introduzione degli alimenti sintetici sul mercato dovrebbe essere quello utilizzato per i farmaci e non certo quello per gli alimenti. Il nostro sistema agroalimentare è un *asset* strategico del Paese. Pensiamo quindi ai milioni di posti di lavoro da preservare, che significano anche un *know-how* importante e prezioso, che non deve essere disperso, ma piuttosto tramandato e conservato, proprio per il suo potenziale di sviluppo, perché rappresenta la nostra cultura e nutre la nostra economia. Chi fa agricoltura e chi fa allevamento è infatti custode del nostro territorio e svolge un ruolo sociale fondamentale per la preservazione delle aree rurali, contribuendo a limitare il dissesto idrogeologico, con quanto ne consegue, specialmente in termini di spopolamento e di abbandono delle campagne. Voglio approfittare di questo provvedimento per sfatare quello che ormai sembra un luogo comune e cioè che l'agricoltura e la zootecnia inquinano. Meglio di noi nessuno può dirlo, perché già dalle prime azioni di governo l'abbiamo dimostrato. Voglio ricordare a tutti l'approvazione della norma sull'istituzione del registro dei crediti di carbonio agroforestali. Ci siamo proposti di conseguire la neutralità climatica entro il 2030

che favoriscono il sequestro del carbonio dei suoli. Non da ultimo, ricordo a tutti l'approvazione della norma che consente la sperimentazione in campo aperto di produzioni ottenute mediante le tecniche di evoluzione assistita, che sono in grado di darci vegetali più resistenti al cambiamento climatico, con minore necessità idrica e con minore utilizzo di fitofarmaci e pesticidi. Per tutto questo rifiutiamo le motivazioni ufficiali a favore della produzione del cibo sintetico. Faccio una mia considerazione, che immagino sia condivisa da parecchi di voi. Penso fortemente che questa proposta, quella della produzione del cibo sintetico, sia la frontiera di un nuovo *business*, intravisto da quelle poche multinazionali che possono permettersi una partita che richiede investimenti e che vale miliardi di euro. A fronte di questo, siamo ancora più motivati a difendere il nostro sistema agroalimentare e il nostro cibo *made in Italy*, che rappresenta la nostra identità e che mai sarà compatibile con la produzione di cibo da un macchinario che si chiama bioreattore.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare riteniamo sia innanzitutto di dubbia utilità e necessità. Anzi, diciamo pure che l'utilità e la necessità sono ancora tutte da dimostrare. La logica che riscontriamo in questo atto segue un po' quella della riserva indiana, Presidente, di chiusura, di protezione sterile, di non scelta o di proibizione aprioristica. un approccio che abbiamo visto per le adozioni monogenitoriali e che vediamo nell'atteggiamento di protezione non ragionata nell'applicazione della direttiva Bolkestein; lo vediamo addirittura in materia di cambiamento climatico. Si vogliono risolvere i problemi non affrontandoli o negandoli, con un *mix* di burocrazia difensiva o addirittura con la rimozione. Il provvedimento risulta figlio di un'impostazione logica pregiudiziale, miope e provvisoria; e vi spiego perché. logica è pregiudiziale perché l'intero impianto del disegno di legge ruota attorno a una concezione non supportata da alcuna base scientifica. Infatti, quando viene richiamato il principio di precauzione per giustificare un'eventuale limitazione della circolazione degli alimenti e dei mangimi a base cellulare, non si tiene conto del fatto che lo stesso principio di precauzione dev'essere preceduto da una valutazione delle informazioni disponibili da cui derivi la possibilità di effetti dannosi per la salute. In questo caso, non essendo pervenuta alcuna valutazione - e lo sottolineo - ufficiale e scientificamente rilevante delle informazioni disponibili, più che di precauzione, si dovrebbe parlare di pregiudizio del Governo su un tema ancora sconosciuto. *(Applausi)*. E arrivo alla miopia con la quale è stata affrontata una tematica che per sua natura esula dai confini nazionali di uno Stato e dai tentativi di regolazione. Con questo disegno di legge si è cercato di imbrigliare e ostruire un tema di cui si sa poco o quasi nulla, talmente sconosciuto che si dovrebbe parlare di ricerca, ancor prima che di divieto. Nel disegno di legge, però, non c'è alcun riferimento alla ricerca; questo vuoto è stato rilevato anche da diversi auditi. Praticamente abbiamo la seguente situazione: il Parlamento si trova a deliberare su un tema non sufficientemente conosciuto e cosa fa, Presidente? Sceglie la strada difensiva, sceglie lo *stop* pregiudiziale e il divieto facile, che non impegna, non sceglie, impedisce ad altri di impegnarsi e sposta in avanti la decisione. Ci saremmo aspettati una scelta diversa, quella della creazione delle condizioni per favorire migliori decisioni future su basi di maggiore conoscenza. Questo come lo si ottiene? Lo si ottiene favorendo e incentivando la ricerca. E invece la si vieta, senza neanche citare la necessità di avviare un percorso di ricerca. In assenza di una disposizione espressa, l'attuale dicitura dell'articolo 2 potrebbe creare problematiche in materia di ricerca o quantomeno scoraggiare le attività di ricerca medesime. Ho definito il provvedimento anche provvisorio, perché gli effetti che questo disegno di legge si accinge a produrre sono destinati a cessare nella misura in cui il settore delle carni e dei mangimi a base cellulare verrà disciplinato dalla normativa europea. Infatti, sebbene il divieto di cui all'articolo 2 venga istituito sulla base del principio di precauzione, desidero ricordare che, qualora un altro Stato membro dell'Unione europea preveda la commercializzazione della carne coltivata, il divieto di importazione sancito dall'articolo 2 del disegno di legge in esame si scontrerebbe con l'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che tutela la libera circolazione delle merci. intervento condividendo una riflessione su quelle che sono le vere ragioni alla base del disegno di legge in esame. Il ministro Lollobrigida, e con lui tutta la maggioranza, ha giustificato l'intervento in materia con la necessità di tutelare, da un lato, dall'*italian sounding* e, dall'altro, di difendere gli agricoltori e gli allevatori italiani. in discussione non ha nulla a che vedere con l'*italian sounding,* che è un problema serio e che necessita di politiche dedicate. Se si vuole affrontare il problema, gli avversari (quelli veri) sono facilmente individuabili nel mercato, di certo non nella carne a base cellulare, che un mercato ancora non ce l'ha. Non ha senso, come non lo ha provare ad aizzare il mondo agricolo, polarizzando così il dibattito ad arte. Le carni e i mangimi da colture cellulari non sono mai stati e mai saranno un'alternativa ai prodotti agricoli di qualità, soprattutto quelli che derivano dalla piccola e media impresa del settore agricolo, che costituiscono la la maggior parte degli operatori del settore agroalimentare. Semmai, questi prodotti possono essere delle alternative (comunque alternative) rispetto alla grande produzione agroalimentare, costituita da multinazionali e non dai nostri agricoltori o dai nostri allevatori. In conclusione, signora Presidente, chiedo per il suo tramite alla maggioranza di valutare in maniera lucida e non strumentale il provvedimento in esame, pensando a quale sarà il ruolo dell'Italia nel settore della ricerca e a quali sono le vere categorie che beneficeranno di questo divieto: non gli agricoltori italiani, le grandi multinazionali. il fatto che l'Italia sia il Paese più bello del mondo non è un'opinione: abbiamo 53 siti UNESCO, siamo numeri uno al mondo, il 70 per cento del patrimonio artistico della terra e una varietà di specie vegetali e animali che ci invidia tutto il mondo. Per quanto riguarda poi la fauna, in Italia abbiamo 58.000 diverse specie, il più alto numero in Europa. Tutto questo e non solo è patrimonio del nostro Paese ed è per questo che come maggioranza siamo particolarmente orgogliosi di aver lavorato al provvedimento in oggetto, che è un chiaro indirizzo politico, così come è altrettanto vero che risulta particolarmente inquietante

che i senatori della Lega Gianmarco Centinaio e Giorgio Maria Bergesio hanno voluto un emendamento, che è stato approvato, affinché entrasse in vigore il divieto di utilizzo di nomi che fanno riferimento alla carne e ai suoi derivati per prodotti trasformati, che invece contengono esclusivamente proteine vegetali. Con l'approvazione di tale emendamento si assicura non solo il diritto dei cittadini a ricevere un'informazione corretta per tutelare la loro salute e i loro interessi, ma si riconosce e si difende anche il valore culturale, socioeconomico e ambientale dei prodotti zootecnici e delle imprese produttrici. Per intenderci, la mortadella vegana non è una mortadella; la bistecca sintetica non è una bistecca. Fate tutte le porcherie che volete, ma non avete il diritto di confondere né di infangare prodotti di eccellenza. Tra l'altro, non è giusto che quella sintetica venga chiamata carne, anche perché non ci sono ancora studi e sperimentazioni credibili sul suo effetto innocuo. Purtroppo, complice la cara Bruxelles,

Si usa genericamente il tema dei Paesi poveri per imporre la ricetta del cuciniere del mondo, condita oggi da parole come *green, food for future*, sostenibilità, ambiente: espressioni di un ideologismo esasperato. I popoli, si sa, si soggiogano con la dipendenza dal cibo e la possibilità di accedere all'acqua. Un certo ambientalismo spinto sulle nostre tavole può essere un cavallo di Troia, ma noi per questo siamo qui e ci saremo ancora. In altre parole, il rischio dello Stato etico, che, con la scusa dell'ambiente, decide la nostra dieta c'è e con questo disegno di legge abbiamo iniziato a fermarlo. Non è un dettaglio che una delle tematiche al centro del *forum* di Davos, come sempre, sia la cosiddetta transizione energetica, nella prospettiva di vincere la sfida rappresentata dal preteso cambiamento climatico di origine antropica. social e governance* (ESG) che orienteranno investimenti pubblici e privati per molti anni a venire, le ultime novità riguardano la transizione alimentare: abbandono degli allevamenti intensivi nella prospettiva del vegetarianismo, dell'introduzione della carne sintetica e degli insetti nell'alimentazione umana. No, signori, Davos non può e non deve imporci alcun decalogo sulla sostenibilità alimentare. *(Applausi)*. Il World economic forum, quello del grande *reset*, ha pubblicato un articolo che riferisce di uno studio psicologico che che analizza i motivi per i quali le persone sono restie a cibarsi di blatte e larve e continuano a preferire costate alla fiorentina, *tartare* al coltello, genovesi, parmigiane di melanzane e sartù di riso. Secondo i filosofi del World economic forum, le suddette preferenze sono semplicemente abitudini culturalmente condizionate, che possono essere modificate nel tempo, utilizzando la parola magica «naturale». In questo modo, sostengono i suddetti filosofi, si può convincere la gente a bere anche acqua di fogna al posto di acqua potabile, ed è proprio ciò di cui parlerò, ma non inquietiamoci. Vi ricordate Bill Gates, il filantropo che si è messo a bere acqua ricavata da feci umane? Allora non vi spaventerete per un poco di acqua di fogna, vero? Non ci pensate al pianeta che avete contribuito a rovinare? Non vorrete mica fare gli schizzinosi. Mi viene in mente il progetto dell'Olanda. Mentre Bruxelles ha stanziato milioni di euro per la ricerca su carne sintetica e proteine alternative per spingere la riduzione del consumo di prodotti di origine animale, l'Italia è la prima Nazione al mondo a vietare la produzione del cibo sintetico. In conclusione, signor Presidente, il nostro Paese chiude quindi le porte a ogni tipo di sperimentazione alimentare, bloccando sul nascere qualsiasi contaminazione che possa arrivare dall'esterno. Il Sud Europa si distingue per biodiversità, come pure per cibi tradizionali che si caratterizzano per il legame con il territorio, ed è quello che il mondo ci invidia. Dall'Italia arrivano i cibi più richiesti. Le recenti classifiche della guida «TasteAtlas» ci collocano al primo posto nel mondo e invece ci vogliono portare, giorno dopo giorno, verso

come cambiamo il modo in cui le persone pensano e parlano di questo? E perché persone adulte, in teoria intelligenti, ignorano la scienza, la matematica e la fisica e non fanno ciò che si dovrebbe fare? È davvero straordinario che noi, una selezione ristretta di essere umani, siamo in grado di sedere in una stanza, trovarci

È iscritta a parlare la senatrice Licheri voglio iniziare questo mio intervento con un ringraziamento a tutto il Governo Meloni, in particolare ai ministri Schillaci e Lollobrigida, per questo provvedimento, che pone l'Italia all'avanguardia, sia nella tutela dei consumatori, sia in tema di difesa delle eccellenze.

un provvedimento del quale è stato detto tutto e il contrario di tutto e sul quale si è creata una mistificazione ingiusta rispetto a un provvedimento che invece guarda alla tutela dei cittadini e dei consumatori. Direi che è unanimemente riconosciuto che le nostre produzioni agroalimentari siano un'eccellenza e che la dieta mediterranea, che si basa proprio sulle nostre produzioni, sia sinonimo non solo di qualità, ma anche di benessere e che la cucina italiana nel mondo non è solo la più apprezzata, tanto che il Governo l'ha candidata ad entrare nel patrimonio UNESCO, ma è anche sinonimo di riconoscibilità del valore delle nostre tradizioni. È una reputazione, quella del *made in Italy* e della produzione di qualità, che è stata costruita nei secoli, frutto del lavoro e della dedizione di tanti, ed è anche una parte imprescindibile di quel *made in Italy* che è sinonimo di qualità in tutto il mondo e che ci rende riconoscibili come marchio di qualità, qualsiasi cosa l'Italia produca. È un patrimonio, quello dell'agroalimentare, quello delle tradizioni e quello dell'allevamento e dell'agricoltura, che il Governo ha scelto di tutelare, di difendere e di valorizzare, attraverso molte azioni

Il disegno di legge che oggi stiamo discutendo e che andrà in approvazione nelle prossime ore vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi cosiddetti sintetici,

con la denominazione di carne, di prodotti che sono trasformati e che contengono esclusivamente proteine vegetali. Con queste azioni si dà attuazione al principio di precauzione previsto dall'Unione europea per la salute dei consumatori e al principio di trasparenza, che ci impone di fornire tutte le corrette informazioni sul cibo, in modo da consentire al consumatore una scelta consapevole e in sicurezza, un po' come è avvenuto anche con la farina di grilli. Secondo gli esperti che hanno sollevato un potenziale problema di sicurezza alimentare, i rischi potrebbero riguardare la trasmissione di patologie dagli animali, che potrebbero derivare anche dall'utilizzo, ad esempio, di ormoni o di altri prodotti chimici che vengono utilizzati per la produzione o il miglioramento di questo prodotto sintetico all'interno dei bioreattori. Processi complessi e complicati, li abbiamo sentiti anche negli approfondimenti, che rendono questi procedimenti più simili a quelli della produzione di farmaci, piuttosto che a quelli alimentari e a questa sfera andrebbero riferiti. Con questo provvedimento, oltre alla salute, la cui tutela dev'essere un pilastro nell'azione di ogni governo e di ogni buon legislatore, si interviene anche a tutelare un sistema produttivo di qualità come quello degli allevamenti e delle produzioni italiani. Ricordiamoci che la grandezza italiana è fatta dalle nostre differenze, dalle peculiarità delle nostre produzioni, dalle particolarità dai piccoli prodotti che non si riesce a copiare, perché sono frutto di una tradizione secolare, che molti ci invidiano e che per questo probabilmente vorrebbero annullare. Il Governo si impegna in questa direzione, e non solo per promuovere il frutto frutto della cultura e dell'ingegno della nostra Nazione, ma anche perché dietro queste volontà e produzioni è ormai molto probabile, se non certo, che ci sia una volontà speculativa ed economica che muove certe scelte; volontà che ci vorrebbe tutti come consumatori appiattiti e omologati, incapaci di scegliere per la qualità, con un prodotto unico offerto attraverso uno scollamento del legame forte fra la terra e le radici dei nostri prodotti e della nostra cultura un qualcosa che viene costruito in laboratorio, lontano dalla natura, dalla nostra tradizione, dalla realtà quotidiana che è stata la crescita economica e fondamentale dell'Italia. La tutela del patrimonio zootecnico nazionale - lo ricordava anche una collega intervenuta prima - è frutto anche di una mobilitazione popolare, di una di una petizione firmata da oltre 1,5 milioni di cittadini italiani, da tanti consigli comunali e regionali che si sono espressi in questo senso, chiedendo al Governo di intervenire

agroalimentare, che sono un'ossatura, non solo storica, economica e culturale, ma anche delle nostre tradizioni.

Diciamo sì alle produzioni di qualità, diciamo sì alla tutela dei nostri consumatori e alla chiarezza verso il consumatore, che deve sapere che cosa va a comprare e che cosa mette sulla sua tavola. Non siamo per i prodotti standardizzati: vogliamo che le persone abbiano la capacità di scegliere liberamente per la loro tutela e per la qualità di ciò che mettono in tavola. Diciamo no a chi vuole trasformare il consumatore in qualcosa di standardizzato, anch'esso in un prodotto dell'omologazione, che ci deve vedere uguali, sia nella produzione che poi nel consumo.

due cose: innanzitutto, i nostri agricoltori e allevatori sono un punto di riferimento preciso e chiaro di tutela del nostro patrimonio ambientale *(Applausi)*. che tradizionalmente mettono nelle realtà che gestiscono, molte situazioni di un territorio già fragile per la condizione ambientale sarebbero drammatiche. Infine, voglio sfatare la questione ambientale, perché i bioreattori consumerebbero molto più di molti degli allevamenti tradizionali che popolano i nostri bellissimi territori. Concludo, signor

troppe volte abbiamo visto spingere avanti le dinamiche legate al mercato economico per accorgersi troppo tardi che certi prodotti avevano fatto troppe vittime sul nostro territorio.

di dipanare la cortina di fumo che ammanta la materia in oggetto; sì, Presidente, perché sul presente disegno di legge governativo, che reca divieti sulla produzione e commercializzazione di carni coltivate, di fumo ce n'è tanto, di arrosto quasi nulla. È un provvedimento ritenuto da una parte della comunità scientifica economicamente, scientificamente e culturalmente insensato, poiché si vieta ciò che è già vietato, che ancora si sta studiando e che potrebbe di fatto rappresentare una grande opportunità per il Paese. È un disegno di legge proibizionista e liberticida, che non presenta uguali in altri Paesi. proibizionista perché, in nome e in difesa del *made in Italy* si proibiscono preventivamente prodotti a base di carne coltivata, che ancora sono in fase di studio e per i quali ancora non è stata presentata alcuna richiesta di approvazione all'Agenzia per la sicurezza alimentare. Presidente, noi tutti siamo per la difesa del *made in Italy*, ma ciò che non si comprende è cosa si debba difendere, visto che l'Italia importa quasi il 50 per cento del suo fabbisogno di carne. Non è vero invece che così si preclude la possibilità di creare filiere di produzione di carne coltivata *made in Italy*? È liberticida perché non si lascia la libertà di scelta ai consumatori, che potrebbero ad ogni modo ritrovarsi comunque sugli scaffali la carne coltivata, prodotta però in altri Paesi dell'Unione europea. Ebbene sì, questo è il rischio per gli italiani. Ad oggi in Europa sono vietate la produzione e la commercializzazione di carne coltivata, perché - come tutti i *novel food* - sono soggetti ad una valutazione del rischio condotta dall'Agenzia per la sicurezza alimentare, che ne dà il nullaosta solo se accerta che il profilo nutrizionale e quello di rischio sono analoghi rispetto ai prodotti che vanno ad affiancare e, solo in caso di positività, la Commissione europea ne autorizza il commercio. A quel punto niente potrà bloccare questi prodotti dall'attraversare le frontiere e arrivare sulle nostre tavole. Qui, Presidente, viene meno anche l'altro argomento che abbiamo sentito avanzare dai presentatori in questi giorni su questo disegno di legge governativo, cioè che si vuole garantire la tutela dei consumatori, mentre è evidente che le cellule staminali necessarie per la produzione di carne colturale sono le stesse che nell'animale compongono alcuni dei tessuti che poi formano una bistecca; cellule appartenenti alla stessa famiglia di quelle che si usano già da molti anni in ambito clinico. Insomma, Presidente, è del tutto evidente che il disegno di legge in esame rappresenta l'ulteriore manifesto ideologico di questo Governo, che pure non sembra mancare di taluni problemi interni da risolvere. A dimostrazione di quanto detto, si evidenzia che i vincoli del presente disegno di legge si applicano solo per gli animali vertebrati e non per la carne coltivata di molluschi, cefalopodi o crostacei. Insomma, carne no, pesce sì. Dunque, Presidente, quello che noi abbiamo chiesto nei lavori di Commissione con i nostri emendamenti era quantomeno di poter salvaguardare tutte le condizioni che permettevano alla ricerca privata italiana di partecipare alla fase importante di nuovi fonti di sostentamento e a quel processo di sostenibilità ambientale che vede l'abolizione di tutte le forme di allevamento non ecosostenibili ed ecocompatibili.

difendere il *made in Italy*, difendere i nostri agricoltori, difendere i prodotti della nostra terra: è la nostra missione, perché un Paese senza agricoltura è un Paese che non ha futuro. La battaglia contro il cibo sintetico è prima di tutto una battaglia di civiltà, di rispetto e di amore per la nostra terra e per il patrimonio agroalimentare italiano, che è sinonimo di cultura, di tradizione e di identità per il popolo italiano. Il disegno di legge presentato dal Governo di centrodestra, che abbiamo migliorato con importanti modifiche in Commissione, è un provvedimento coraggioso che farà dell'Italia il primo Paese al mondo a vietare il cibo sintetico Quella contro il cibo sintetico è una battaglia che la Lega ha iniziato, per prima e da sola, molti anni fa nel silenzio generale della politica italiana ed europea, fin da quando nel lontano 2013 - quindi dieci anni fa - nella mia veste di europarlamentare avevo denunciato alla Commissione europea la follia del primo *hamburger* sintetico *(Applausi)*, prodotto in Olanda per la modica cifra di 325.000 dollari. Ancora una volta, quindi, i fatti hanno dimostrato che avevamo ragione noi, che per primi avevamo compreso la pericolosità dell'operazione cibo sintetico. Da anni, infatti, il *made in Italy* e l'agricoltura italiana sono diventate oggetto di attacchi furibondi da parte delle *lobby* e delle multinazionali del cibo sintetico; attacchi portati avanti con la colpevole complicità dell'Europa, che in questi anni ha sostenuto e persino finanziato la produzione del cibo sintetico. È chiaro a tutti, ad eccezione della sinistra *radical chic*, che la produzione e la diffusione su vasta scala di questi cibi sintetici rappresenta un pericolo mortale per tutto il settore agroalimentare italiano. Il caso più conosciuto è sicuramente quello della carne sintetica, la famosa carne finta fatta in laboratorio, al cui interno non c'è un solo milligrammo di carne. Com'è possibile spacciare e vendere come carne prodotti che non contengono la minima traccia di carne? I consumatori e gli allevatori italiani vanno tutelati, non truffati per compiacere gli interessi delle multinazionali. Proprio per questo, grazie a un emendamento della Lega, l'articolo 3 del disegno di legge vieta espressamente anche l'uso fraudolento della denominazione «carne» e dei termini che richiamano la carne abbinati a questi prodotti. Il fenomeno del cibo sintetico, che sta pericolosamente prendendo piede in Europa, non riguarda però soltanto la carne. Per tali motivi, con il disegno di legge in discussione diciamo un no forte e chiaro a tutti gli alimenti e a tutti i mangimi sintetici: no al latte sintetico (il famoso latte senza le mucche); no ai formaggi senza latte; no al pesce sintetico prodotto in laboratorio. Permettetemi di allargare il ragionamento. La Lega dice di no anche a tutte le altre follie alle quali Bruxelles vuole spalancare le porte: no al vino senza uva; no al vino senza alcol; no a vermi, insetti e cavallette, che i burocrati europei vorrebbero portare sulle tavole degli italiani. È evidente a tutti che il cibo sintetico fa parte di un disegno più generale, insieme al Nutri-score e alla strategia *farm to fork*, con il quale l'Europa punta a scardinare il modello agricolo e alimentare del *made in Italy*. Ben venga allora questo disegno di legge, che passerà alla storia per essere il primo provvedimento legislativo al mondo che vieta la produzione, l'utilizzo, l'importazione e la vendita di prodotti realizzati in vitro, raccogliendo in questo modo l'appello arrivato da 2.000 Comuni, dalle Regioni, da migliaia di cittadini e dalle imprese del settore agroalimentare, che valgono la bellezza di 522 miliardi di euro, pari al 15 per cento dei PIL italiano. Il valore di questa legge è anche e soprattutto di natura politica, perché con essa mandiamo un messaggio politicamente molto forte - ripeto, molto forte - a Bruxelles, dove si decidono le sorti dell'agricoltura italiana ed europea. Noi italiani non molleremo di un centimetro nella battaglia per difendere il *made in Italy*, che rappresenta un patrimonio unico al mondo fatto di qualità, tipicità e legame con il territorio. I burocratici di Bruxelles si mettano l'anima in pace. La Lega, il Governo di centrodestra, noi italiani siamo pronti a lottare con ogni mezzo per difendere la nostra sovranità alimentare e il patrimonio agroalimentare del nostro meraviglioso Paese. Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli sarò estremamente sintetico e utilizzerò molti meno minuti di quelli a disposizione, perché ho avuto modo di ascoltare con grande attenzione l'intervento della relatrice Cantù e dei colleghi del mio Gruppo parlamentare, Leonardi e Nocco, che hanno esternato in maniera ineccepibile ed esaustiva alcune riflessioni, che sottoscrivo in pieno. Ci tengo però a fare alcune brevi riflessioni in merito al disegno di legge in esame che - come è stato ampiamente detto propone di vietare la produzione, la commercializzazione e l'importazione della carne coltivata. Si tratta di una legge che è stata fortemente voluta dai ministri Lollobrigida e Schillaci, ma che è stata anche sollecitata da 1.200.000 italiani, che hanno sottoscritto una petizione di Coldiretti. È stata altresì sollecitata da 3.150 Consigli comunali, che hanno approvato un ordine del giorno in tal senso, e da quasi tutti i Consigli regionali della nostra Nazione. una norma che applica il principio di precauzione, inserito all'interno del Regolamento n. 178 del 2002, precisamente all'articolo 7, in riferimento a situazioni di incertezza sul piano scientifico, che ha un obiettivo prioritario: quello della tutela della salute pubblica. Si tratta di un obiettivo di fondamentale importanza, come lo è certamente un altro obiettivo perseguito da questo disegno di legge, ovvero la tutela del nostro patrimonio agroalimentare, che è sinonimo di qualità e che è anche un modo attraverso il quale si esprime la nostra identità culturale. un patrimonio agroalimentare sinonimo di qualità, invidiato da tutto il mondo. Se è vero, come è vero, che l'Italia è la Nazione al mondo con il più alto numero di prodotti DOP, IGP e STG,

metterebbe a rischio milioni di posti di lavoro, laddove certamente poche multinazionali andrebbero a produrre cibi sintetici, andando a delocalizzare le proprie produzioni all'interno di altri contesti territoriali, dove il costo del lavoro è certamente inferiore. Si determinerebbe altresì l'abbandono di intere aree extraurbane della nostra Nazione, con conseguenze disastrose anche dal punto di vista ambientale. Soprattutto - come è stato detto da molti colleghi che si sono alternati prima di me - i cibi standardizzati andrebbero a eliminare il concetto di qualità, che rappresenta un elemento qualificante della nostra Nazione, di cui tutti dobbiamo essere assolutamente orgogliosi. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, ci troviamo a discutere in quest'Aula l'ennesimo provvedimento governativo che, coerentemente con gli intenti oscurantisti dei suoi proponenti, dimostra di voler osteggiare e frenare la crescita e lo sviluppo scientifico, ambientale ed economico del Paese. Siamo infatti dinanzi a un progetto di legge figlio di una logica politica bigotta e conservatrice, fondata sull'idea di repressione quale unico strumento per fronteggiare le trasformazioni e le evoluzioni che investono la nostra società civile. Nella fattispecie, oggi dibatteremo sull'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento - leggo testualmente dal titolo del disegno di legge in esame - il «divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici». un divieto che di per sé non ha motivo di essere istituito, dato che ad oggi non si registra alcuna norma, né a livello nazionale né a livello europeo, che regolamenti in Italia la produzione e la commercializzazione della cosiddetta carne sintetica, così erroneamente chiamata. Il termine corretto in uso nella comunità scientifica è infatti quello di «carne coltivata». Con la presentazione di questo testo si è arrivati all'apoteosi dell'atteggiamento proibizionistico e sanzionatorio di questo Governo, il quale, perseguendo le proprie logiche retrograde, si è addirittura spinto a colpire un prodotto non ancora in commercio in Europa. Sin dalla relazione illustrativa, questo provvedimento dimostra di voler criminalizzare preventivamente e immotivatamente una ricerca che potrebbe costruire una delle possibili soluzioni all'insostenibilità del sistema alimentare attuale e, al contempo, contribuire a compensare la grave carenza alimentare presente in vaste aree del nostro pianeta. È imbarazzante e dilettantistica la scelta del Governo di utilizzare in un provvedimento legislativo una terminologia faziosa e scientificamente imprecisa, volta a manipolare il consumatore instillandogli la convinzione che la sperimentazione della carne coltivata sia un prodotto sintetico creato in laboratorio, un cibo finto che rimanda, nell'immaginario collettivo, alla plastica, alla resina o al petrolio e per questo dannoso per la salute. Considerazioni campate per aria, nel cui merito in Commissione purtroppo non si è potuti entrare, dato che di fatto è stata impedita la reale possibilità di instaurare un serio contraddittorio, esautorando l'opposizione del diritto di aprire un fondato fronte di dialogo con la maggioranza. In questa Aula, Presidente, colgo infatti l'occasione per rivolgermi al presidente Zaffini, segnalando come anche da parte sua ci siano stati un muro e l'indisponibilità ad interloquire in merito alla scelta dei soggetti da audire nello svolgimento dell'istruttoria. Oltre a ledere il sacrosanto diritto di rappresentanza di ogni Gruppo parlamentare, non si è voluto dare la giusta voce e il giusto spazio al mondo della scienza e della ricerca, impedendo in tal modo a noi commissari di acquisire un ampio spettro di informazioni su cui incardinare un dibattito costruttivo, aperto ed informato. Tale gestione dei lavori ha inoltre privato il cittadino della possibilità di ascoltare via *streaming* i pareri tecnici delle personalità da noi segnalate. Mai come in questa occasione mi sento di dire di aver assistito a una vera farsa, che ha rivelato anche tutta la fragilità e la debolezza della tesi governativa sulla tematica della carne coltivata. Troppo facile negare il legittimo diritto al contraddittorio, per poi lanciarsi in interpretazioni pindariche sull'argomento. Ma, lasciando da parte le scorrette prassi operative e decisionali di questo Governo, a cui personalmente non mi abituerò mai e che non smetterò mai di evidenziare, ciò che preme a noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra è di illustrare i profili maggiormente critici di questo irragionevole disegno di legge, che, qualora venisse approvato, contribuirebbe ad accrescere l'isolamento dell'Italia rispetto all'opportunità di trasformare la produzione e il consumo di carne anche su scala internazionale. A questo proposito, infatti, è essenziale ricordare come il *green deal* europeo, che rende giuridicamente vincolante l'obiettivo di ridurre le emissioni del 55 per di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, dovrà essere raggiunto con l'aiuto di tutti i settori, compreso quello agroalimentare. In una fase ancora sperimentale rispetto al lancio sul mercato di prodotti a base di cellule coltivate di origine animale, più che vietare l'avvio di qualsiasi studio sull'argomento risulterebbe quanto mai necessario promuovere invece un'attenta e corretta analisi scientifica sulle implicazioni che simili colture potrebbero generare in termini di impatti economici, ambientali e sociali: risparmio di elettricità, di acqua, di antibiotici, di additivi e abbattimento delle emissioni climalteranti. Analisi che andranno necessariamente confrontate con quelle già esistenti, riguardanti le modalità di produzione della carne convenzionale. Si pensi ad esempio agli allevamenti intensivi ed estensivi. In termini comparativi sarà di essenziale importanza verificare quanto la produzione della carne coltivata possa ridurre la quantità dei terreni utilizzati per l'allevamento (i quali potrebbero essere piuttosto oggetto di riforestazione e/o di produzione di altre colture alimentari ambientalmente meno impattanti), l'utilizzo delle risorse idriche, la produzione e la commercializzazione di fertilizzanti dannosi alla salute e all'ambiente, le emissioni di gas connessi allo smaltimento e alla fermentazione dei liquami prodotti dai bovini da macellare. Coniugata alla motivazione ambientale vi è poi una motivazione di matrice economico-sociale: impedire che in Italia vengano sviluppate delle ricerche nel settore dell'agricoltura cellulare penalizzerebbe fortemente il nostro mercato interno, il quale si troverebbe ad essere marginalizzato in un settore che, oltre ad essere in forte espansione nei Paesi europei ed extraeuropei, presenta già da ora enormi potenzialità di crescita sotto il profilo economico e lavorativo. Adottare una politica di apertura su questo tema consentirebbe alle aziende italiane di investire nello studio e nella ricerca, favorendo così la nascita di un nuovo tipo di industria avente delle ricadute positive anche in termini di occupazione al contempo, nuove sperimentazioni nel campo della cosiddetta medicina rigenerativa. È dannoso, oltre che scorretto, fomentare l'idea che l'arrivo sul mercato della carne coltivata soppianti la commercializzazione dei prodotti di eccellenza tradizionalmente prodotti e distribuiti dalle virtuose aziende italiane. È quindi del tutto evidente e logico che il Governo, proibendo questa ricerca, si getterà letteralmente una zappa sui piedi, visto e considerato che in seconda battuta, data la vigenza del diritto della libera circolazione delle merci in territorio europeo, l'Italia sarà costretta ad importare questi prodotti da altri Paesi. In ultimo, l'ulteriore tema da affrontare è quello connesso ai rischi per la salute dei consumatori. legge in esame, infatti, rintraccia la propria *ratio* esattamente nella necessità di tutelare la salute degli esseri umani rispetto agli effetti cancerogeni derivanti dal consumo di alimenti prodotti artificialmente, tra cui la carne coltivata. Si segnala però come questo assunto non abbia delle valide evidenze scientifiche: non le può avere, dato che la carne coltivata non è ancora in commercio. Per contro, sussistono solidi dati scientifici che certificano il rischio per la salute provocato dall'abuso di carne rossa. Senza entrare in tecnicismi, basta riprodurre lo stesso testo presente nella relazione illustrativa del provvedimento per comprendere come lo *status* della ricerca e della sperimentazione degli alimenti coltivati sia in una fase così embrionale tale per cui non si è nelle condizioni di avanzare alcuna ipotesi circa la pericolosità di questi *novel food.* Brevemente, prima di concludere il mio intervento, vorrei inoltre sottolineare la debolezza giuridica e il potenziale profilo di illegittimità discussione andrebbe incontro qualora diventasse legge. Si ricorda, infatti, come il principio di precauzione su cui questo si fonda, mutuato dall'articolo 7 del regolamento della Comunità europea n. 178 del 2002, preveda l'introduzione di misure restrittive al commercio solo ove permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico circa la pericolosità dell'alimento considerato. Superata questa ipotesi di pericolosità, dette misure (e nel nostro caso l'intera impalcatura del disegno di legge oggi in esame) non avrebbero più alcun fondamento giuridico e così di nuovo, invece di concentrarsi sui veri problemi che attanagliano l'Italia, sulle vere priorità di questo Paese, quali la messa in sicurezza del territorio e delle persone che vi abitano, due Commissioni si sono occupate per settimane di un fantomatico prodotto non ancora esistente, con un vero spreco di risorse e di tempo. rappresentanti del Governo, innanzitutto sgombriamo il campo dalle *fake news:* la carne sintetica non esiste e non esisterà mai. La denominazione di carne sintetica è una vera *fake news* che ha tratto in inganno tantissimi cittadini e tantissime istituzioni *(Applausi)*, ma è assolutamente falso il concetto che quel possibile potenziale alimento sia sintetico. In realtà, in vari Paesi del mondo è stata avviata da qualche tempo la ricerca del modo di produrre con un procedimento biochimico un alimento ad alto contenuto di proteine animali, che sono necessarie per l'alimentazione anche in Italia sono partite ricerche di questo tipo, per esempio a Trento e a Tor Vergata. Questo alimento ad alto contenuto di proteine animali deriverebbe, se la ricerca porterà a ottenere un procedimento sostenibile e corretto dal punto di vista igienico-sanitario, dalla moltiplicazione controllata in laboratorio di cellule staminali. di cellule staminali. Per chi non lo ricordasse, le cellule staminali sono le cellule iniziatiche che in tutti gli organismi viventi, moltiplicandosi, fanno sì che l'organismo abbia le diverse cellule che lo compongono. Tutto parte, però, dalle cellule staminali. Quindi, le cellule staminali sono particolarmente preziose e particolarmente ricercate da decenni per vari scopi, in particolare per scopi medici e curativi, e curativi, e verrebbero prelevate in modo del tutto indolore da animali domestici allevati a scopo alimentare. Il prelievo equivale, come modalità, a un prelievo di sangue. È stata definita carne perché il processo biologico per ottenerla è simile a quello che avviene nell'organismo animale, ma potrebbe tranquillamente essere definita in un altro modo. Anzi, sono convinto che sarebbe stato meglio definirla in altro modo, perché ci sono tanti alimenti derivati che hanno nomi diversi da quello di partenza, come il formaggio rispetto al latte o gli insaccati rispetto alla carne da cui provengono. Ovviamente, una eventuale produzione industriale, ammesso che sia possibile, dovrà essere certificata sotto il profilo igienico sanitario, ma ci vorranno anni per scoprirlo. Come paragone, ricordo che il primo trapianto di midollo osseo, oggi abitualmente impiegato per curare i malati di leucemia (anche in

Quindi, vedete come la ricerca abbia bisogno di tempi per arrivare a produrre protocolli accettabili nella nostra società civile, ed è giusto che sia così. La cosa fondamentale, però, è lasciare che la ricerca possa progredire senza ostacoli burocratici. Infatti, come accaduto in tante altre situazioni, essa potrebbe portare scoperte applicabili in altri ambiti, per esempio nel prevenire malattie nuove o conosciute negli animali d'allevamento oppure nell'individuare potenzialità nutritive oggi sconosciute, per esempio con riguardo alle persone affette da intolleranze alimentari. E non diciamo che la ricerca scientifica non è impedita da questo provvedimento. Certo che lo è. è. Lo dimostrano gli Ogm, che in Italia sono vietati. Nessuno li studia e nessuno li produce: è stata una decisione del Paese, ma poi il Paese spende cinque miliardi di euro all'anno per importarli, perché sono fondamentali, soprattutto per alimentare gli animali di allevamento. Allora, se vogliamo continuare sulla strada della dipendenza dagli altri perché vogliamo essere duri e puri, va bene, ma non so quanto questo ci porti avanti nella comunità internazionale. Tra gli argomenti principali che sento ripetere dai promotori della legge c'è la difesa del *made in Italy*. Siamo tutti d'accordo: chi potrebbe non essere d'accordo.

piccoli e fatti crescere in Italia. Quindi, buona parte del prosciutto e del salame italiano viene realizzata con animali che nascono all'estero. Ricordo che l'Olanda ha investito forti somme, sia private che pubbliche, in questo tipo di ricerca ed è un grande fornitore di maiali appena nati all'Italia. Attenzione, dunque, perché potremmo ritrovarci, un domani, a non avere più la materia prima per fare prosciutti *made in Italy*. Forse è il caso di pensarci. Ricordo anche che, cinquant'anni fa, il *made in Italy* alimentare era diverso da oggi e probabilmente sarà diverso tra cinquant'anni. Tutti ricordate il film di De Sica, "Ladri di biciclette", in cui il protagonista porta il figlio in un ristorante a mangiare la mozzarella in carrozza, perché, all'epoca, era il piatto tipico del *made in Italy* a Roma. Oggi dove la trovate più la mozzarella in carrozza a Roma? La trovate, sì, probabilmente, in alcuni locali, ma

non hanno tenuto conto. Alcuni di quegli studiosi hanno potuto parlare in un convegno istituzionale, organizzato dal Gruppo delle Autonomie lo scorso 13 luglio, dove hanno portato una serie di argomenti che dimostra come questo provvedimento sia assolutamente inutile e sproporzionato. Ricordo che il principio di precauzione si è dimostrato, sia nelle relazioni pervenute alle Commissioni sia nel convegno, come assolutamente non fondato. Lo hanno detto i biotecnologi della società italiana di settore; lo ha detto il comandante di divisione dei Nas, Paolo Carra, audito il 21 di giugno; lo ha detto l'EFSA, anche essa in audizione. In sintesi, oggi questa legge è inutile, perché vieta qualcosa che di fatto è già vietato, visto che nessun prodotto a base di carne coltivata ha iniziato l'*iter* di autorizzazione in Europa e quindi non può essere commercializzato. Questa legge sarà inutile, e aggiungo potenzialmente dannosa domani, se e quando EFSA darà il proprio nulla osta ad alcuni di questi prodotti che potranno essere commercializzati in tutta Europa. Infine, faccio alcune considerazioni sugli sugli argomenti a sostegno del primato mondiale italiano del divieto alla carne coltivata: i bioreattori. Per spaventare i cittadini si è detto che la carne coltivata proviene da bioreattori. Ricordo che lo yogurt, la birra e il vino si fanno in contenitori che tecnicamente sono dei bioreattori. di cavie umane. Per spaventare i cittadini si è usato il mantra terroristico delle cavie umane, ma ci si dimentica che le cellule staminali - come detto prima - sono studiate da decenni in Italia, sono state approfondite in tutti

prelevare le cellule staminali per fare questo prodotto, ma si può fare con i non vertebrati. Quindi i divieti di questa legge valgono per i bovini, ma non valgono per i gamberi e le aragoste. Perché? Sarebbe importante che il Governo ce lo spiegasse, perché potrebbe anche succedere che le aragoste e i gamberi prima o poi verranno prodotti nei bioreattori, per cui magari i pescatori di gamberi e di aragoste potrebbero rimetterci. come illustrato sopra, la possibilità di una concorrenza della cosiddetta carne coltivata - ma chiamiamola in un altro modo: sono d'accordo con la senatrice Bizzotto - con la ho visto - debbo dire - analoghe levate di scudi quando i ristoranti vegani iniziarono a vendere *tofu* e *hamburger* vegetali, ma forse quella volta Coldiretti era disattenta. Cito Coldiretti a caso. Signora Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, ho sentito da più parti parlare di protezione del *made in Italy*, rispetto degli agricoltori e degli allevatori, quindi della zootecnia. Ma ci sono diversi modi per tutelare la zootecnia nazionale e il *made in Italy* è il fatto importante. Porre un divieto sugli alimenti derivati da colture cellulari non è il metodo giusto. un divieto strumentale, fittizio che, se non fosse per il fatto che è necessario per distogliere l'attenzione su temi ben più scottanti e soprattutto screditanti a causa dell'attuale Governo, verrebbe da chiedersi se chi lo propone e lo difende debba fare un bel ripasso di legislazione sul *novel food*. Sulla scrivania del presidente Meloni - metaforicamente parlando - ci sono questioni che urlano vendetta: i ritardi vergognosi nell'attuazione del PNRR, le scivolate sulla politica internazionale e sull'interpretazione del fenomeno migratorio, oltre a guai giudiziari di varia natura e gravità, tanto per fare un esempio; e ancora l'emergenza abitativa, i tassi dei mutui alle stelle, i salari al di sotto della soglia del sostentamento, come dimostrano i fatti. detti problemi hanno, nella scala delle priorità di questo Esecutivo, un grado di importanza limitato, sicuramente inferiore a quello dell'introduzione nel mercato italiano di un prodotto che attualmente non è consentito commercializzare. Perché allora impegnarsi a vietare qualcosa che già implicitamente è impossibile consumare? Un disegno di legge voglio ricordare che ha occupato anche un intero consesso di Ministri riuniti in consiglio, quello del 28 marzo scorso, che forse avrebbero fatto meglio a considerare che le urgenze sono ben altre. Abbiamo il dovere di non tarpare le ali alla scienza, di non rinunciare alla modernizzazione. L'Italia non può diventare un Paese retrogrado, coperto dalla polvere dell'oscurantismo e del pregiudizio. La ricerca scientifica è sacra ed è chiaro che, se si pongono divieti aprioristici, si scoraggia qualsiasi forma di approfondimento, analisi e sviluppo, anche perché tra l'altro la ricerca non vive solo di fondi pubblici. Se questo disegno diventerà legge, vorrà dire anche, tra le varie cose, che si darà un ulteriore motivo a tanti giovani di scappare, alimentando quella che è già una grave emorragia italiana: la fuga dei cervelli, delle nostre eccellenze in fatto di ricerca. Nell'anno 2023 - ripeto, 2023 - l'agricoltura fa il paio con l'innovazione tecnologica, con strumenti e tecniche avanzatissime in grado di porre rimedio ai grandi drammi del nostro tempo (il consumo del suolo, l'emergenza climatica, la perdita di biodiversità, il dissesto idrogeologico). Ci domandiamo allora come sia possibile che un partito, quello che conta qui più rappresentanti, possa, da un lato, portare avanti le tecniche di evoluzione assistita nel settore primario - slancio di modernizzazione agricola - e, dall'altro, sempre in campo agricolo, possa vietare uno stesso slancio di modernizzazione. «Dobbiamo fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico e, allo stesso tempo, soddisfare le richieste alimentari di una popolazione mondiale in crescita. Solo migliorando le *performance* e riducendo le necessità in termini di acqua, fertilizzanti e farmaci possiamo affrontare queste sfide», citazione testuale del senatore De Carlo a proposito di tecniche di *editing* genomico, che potrebbero essere adoperate senza battere ciglio anche per gli alimenti colturali che, sottolineo ancora, sono totalmente in linea con le finalità delle Dico questo non per fare delle sovrapposizioni argomentative audaci, ma per dare enfasi ad un concetto molto semplice, a quanto pare poco chiaro a molti presenti, per raggiungere un medesimo obiettivo, in questo caso la salvaguardia del pianeta. Per fare questo ci sono diverse strade, tutte ugualmente valide, specie se si procede per tentativi. Innescare la politica della proibizione e della negazione a tutti i costi non renderà l'Italia un Paese migliore; piuttosto lo confinerà a fanalino di coda nelle classifiche mondiali delle Nazioni che hanno rifiutato aprioristicamente di capire, di innovare, di trovare soluzioni e, soprattutto, di crescere. Anche il veto sulla possibilità di poter definire un cibo a base vegetale *hamburger* di soia o prosciutto *veg* perché dovrebbe confondere chi va a fare la spesa? Questi riferimenti piuttosto aiutano a capire la consistenza del prodotto e il suo aspetto e il suo utilizzo. Un altro concetto importante è supportare il percorso delle alternative proteiche a quelle di origine animale e ciò non significa stroncare gli allevatori: sappiamo bene, infatti, che specie in cucina è il consumatore a veicolare il mercato. La realtà è che chi vorrà concedersi un'ottima fiorentina al sangue continuerà a farlo, chi vorrà mangiare bistecche di tofu continuerà a farlo. Chi vorrà in un'ottica futura provare un *hamburger* di carne colturale lo farà, con buona pace di chi ci vedeva strane distorsioni delle produzioni nazionali. La narrazione di molte grandi associazioni di categoria, oggi purtroppo totalmente asservite alle logiche di chi siede al potere, ha diffuso questo retro-pensiero del tutto tendenzioso. Si tratta però di falsi allarmismi, che non fanno altro che accrescere disinformazione e allargare il circolo vizioso delle paure infondate. Vi sembra che ci sia stato un'invasione di insetti a tavola, dopo il via libera dell'Unione europea alle farine di grilli? Oggi si possono acquistare, ma non mi pare che le industrie dei prodotti convenzionali da forno ne abbiano risentito. Chi a colazione mangia fette biscottate di farina integrale al 100 per cento italiana, con un velo di miele bio, anche questo totalmente prodotto in Italia, continuerà a farlo e non sarà certo un salatino con farina di grillo posto nella vetrina di qualche negozio a turbare i suoi pasti. Detto questo voglio confermare, se ancora non fosse sufficientemente chiaro, il totale sostegno del MoVimento 5 Stelle al mondo allevatoriale anche in questa sede, dalla ripresentazione degli emendamenti sul rifinanziamento del Fondo nazionale per la suinicoltura e sul fondo degli allevamenti sostenibili. Chi dice il contrario vuole portarvi fuori rotta. Ci tengo a ribadirlo in maniera diretta ai tanti allevatori che ho avuto occasione di ascoltare e incontrare in questi anni. Concludo, signor Presidente, con una rassicurazione per tutti gli operatori della filiera agricola. Noi ci siamo e ci saremo sempre. L'importante è non permettere a strategie distrattive, come quella attuata con la presentazione di questa proposta del tutto superflua, di prendere il sopravvento. Canalizziamo insieme tutte le energie per costruire qualcosa di veramente utile per il nostro magnifico *made in Italy* agroalimentare e per l'agricoltura del futuro.

l'assetto del mondo che è uscito dalla Seconda guerra mondiale: oltre alle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza e alla Corte di giustizia internazionale, abbiamo anche la Corte penale internazionale. Si tratta di una Corte che serve a perseguire reati commessi da singoli individui, reati gravissimi, come il reato di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, il crimine di invasione: tutti reati che fino ad allora non erano perseguiti, se non qualche volta con tribunali *ad hoc*. Ricordiamo ovviamente il processo di Norimberga, o il tribunale che le Nazioni Unite crearono per la guerra nella ex Jugoslavia o in Ruanda. Mancava però un'entità che assicurasse, oltre alla pace, la giustizia. Vede, signora Presidente, la pace non è soltanto la cessazione del risuonare delle armi, non è soltanto ottenere un cessate il fuoco e che in un Paese in guerra si smetta di sparare. La pace si ha quando anche le esigenze di giustizia vengono soddisfatte e quando chi ha utilizzato la guerra per per compiere reati orribili viene assicurato alla giustizia; ancor meglio, viene assicurato alla giustizia, grazie alla Corte penale internazionale, non soltanto dal Paese nel quale il reato è stato commesso, ma dall'intera comunità internazionale. Io voglio ricordare che l'ultimo mandato di cattura della Corte penale internazionale è stato proprio nei confronti di Vladimir Putin e della commissaria russa per l'infanzia per la deportazione di centinaia, forse migliaia di bambini dall'Ucraina. Questo ci dà il senso non soltanto di quanto orribile sia quella guerra, ma anche di quanto sia sbagliato e violento l'atteggiamento con il quale Vladimir Putin ha ordinato l'aggressione nei confronti dell'Ucraina. Con la ministra Cartabia nel marzo del 2022 si era costituita una Commissione, presieduta da due importanti giuristi, i professori Palazzo e Pocar, che doveva servire ad allineare il nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale. Purtroppo, questo Governo non sta dando seguito al lavoro di quella Commissione. Quindi, vorrei formalmente invitare il ministro Nordio e la presidente Meloni a dar seguito a quel lavoro e allineare il nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale. Da ultimo, parliamo di giustizia internazionale e non possiamo non pensare alla sentenza vergognosa che oggi un tribunale egiziano ha emesso emesso nei confronti di Patrick Zaki, condannato a tre anni. Penso che questa sia un'ulteriore lesione, oltre che del diritto, della ragionevolezza e di ogni principio democratico, anche dei buoni rapporti che intercorrerebbero

Signora Presidente, intervengo anch'io su questa giornata importante e sulla Corte penale internazionale.

quello che è fondamentale per questo istituto, cioè lo Statuto della Corte penale internazionale, nel quale sono contenute le norme e le modalità di applicazione di un principio importantissimo. principio importantissimo. Quando parliamo di crimini di guerra, di crimini di contro l'umanità, di aggressioni di Stati nei confronti di altri Stati, rientriamo nel concetto generale di diritti umani. umani, in quanto universali, devono preesistere a qualsiasi altra forma di diritto o di legge e quindi vengono prima delle leggi. Attenzione, i diritti umani preesistono alle leggi

dei Paesi che vi si riconoscono. L'altra strada da percorrere è quella del grande supporto nella raccolta delle prove per questi crimini internazionali. Voglio citare

dal nostro attuale Ministro della giustizia. Le ragioni che sono infatti alla base di questo istituto stanno in quell'impostazione tutta crociana che vede la storia come una storia delle idee e delle libertà. Voglio ricordare una prolusione che fece Giuliano Vassalli nel lontano 1946, quando ricordò e illustrò quanto fosse suggestivo per le nuove generazioni

È un istituto della pace e deve essere un qualcosa che preesiste nelle relazioni internazionali. Cito anch'io la vergognosa questione

Questo rispetto non può e non deve piegarsi a nessuna ragione, né di rapporti internazionali né di qualsivoglia ragione. Questo è un grande passo nella modernità della storia, nella tradizione delle migliori garanzie, nella tradizione delle democrazie liberali. Credo che noi su questo dobbiamo insistere per dare un grande contributo e oggi fare in modo che il Governo italiano prenda posizione e faccia sentire la sua voce con l'Egitto. *(Applausi)*.

sono i giorni che hanno separato le uccisioni dei due magistrati antimafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e che li hanno uniti per sempre nella morte e nell'immaginario collettivo come due eroi a presidio della legalità nella lotta contro la mafia. giorni. Paolo Borsellino era preoccupato per la sua famiglia e per gli uomini della scorta. Chiese più volte agli organi competenti di bonificare i luoghi che frequentava abitualmente; in particolare, chiese la rimozione delle auto parcheggiate in Via D'Amelio, dove si recava spesso in visita alla madre. giorni, ma nessuno fece nulla. Sarebbe bastato forse un divieto di sosta e invece le auto della scorta dovevano impegnarsi in lunghe e lente manovre che hanno reso sin troppo semplici l'agguato e la strage. Era il 19 luglio 1992 e domani se ne celebrerà la ricorrenza. Nella voragine di sangue lasciata dall'esplosione, la madre di Borsellino ha posato una piantina di ulivo, proveniente da Betlemme: l'ulivo, la pianta perenne, l'albero simbolo di pace e di rigenerazione. Da allora sono trascorsi ormai trentuno anni. Oggi quella piantina è cresciuta e sfoggia una meravigliosa ampia chioma, che accoglie ogni giorno il pellegrinaggio di chi conserva nel cuore la gratitudine verso quel giudice coraggioso e determinato sino alla morte e il riconoscimento al valore del suo instancabile lavoro. Ma ancora, purtroppo, quel luogo della memoria è soffocato, oggi come allora, tra le auto parcheggiate. Salvatore Borsellino, il fratello del giudice, che da sempre ne coltiva la memoria, ha recentemente avviato una petizione popolare che ha già raccolto decine di migliaia di sottoscrizioni, tra cui la mia, per la realizzazione in via D'Amelio del Giardino della memoria e per la declaratoria di monumentalità dell'ulivo. Il Comune di Palermo ha accolto la sollecitazione, emanando un atto di indirizzo. L'auspicio di tutti è che le enunciazioni si trasformino presto in fatti concreti e su questo vigilerò, perché iniziative come questa hanno un potente valore simbolico e la rigenerazione urbana diventa simbolo di rigenerazione delle coscienze. È importante che le istituzioni non abbassino la guardia e si mantenga vivo il ricordo del sacrificio di chi ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato e alla lotta contro quella forma di diffusa illegalità che è la mafia. Auspico che tutte le istituzioni si associno al sostegno dell'iniziativa di Salvatore Borsellino, per la creazione del Giardino della memoria, per donare ai pellegrini un luogo consono al raccoglimento e per restituire a quel luogo la sacralità che merita.

legge:"Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano" (755) (presentato